L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.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 Onorevoli colleghi, come è tristemente noto, nella notte del 22 luglio scorso il crollo improvviso di un ballatoio al terzo piano dello stabile popolare Vela Celeste, nel quartiere di Scampia a Napoli, ha provocato due vittime e 13 feriti, tra cui sette bambini di età compresa tra i due e i dieci anni, purtroppo in condizioni gravi o gravissime. Il crollo ha inoltre comportato la necessità di evacuare circa 800 persone, di cui 300 minori, per consentire le necessarie verifiche tecniche sull'edificio, e molti non potranno rientrare a breve nelle proprie case, viste le condizioni dello stabile. Le cause e la dinamica di questo disastroso crollo saranno - come è necessario - oggetto di indagini da parte delle autorità competenti. Desidero, in questa sede, esprimere a mio nome personale e di tutta l'Assemblea sentimenti di cordoglio alle famiglie delle vittime, di vicinanza e incoraggiamento ai numerosi feriti e ai loro cari, nonché di partecipe solidarietà agli sfollati. Sono certa, inoltre, di dare voce al sentimento di tutti i colleghi senatori nel rivolgere un commosso ringraziamento a quanti si sono prodigati nell'emergenza, dai Vigili del fuoco agli operatori della Protezione civile, dalle Forze dell'ordine al personale dei servizi sanitari e ai tanti cittadini accorsi spontaneamente per prestare aiuto. In segno di cordoglio per le vittime di questo gravissimo incidente, invito i colleghi a osservare un momento di raccoglimento.

Signor Presidente, colleghi senatori, tra pochi giorni, il 28 luglio, si terranno in Venezuela le elezioni per scegliere il Presidente che dovrà guidare il Paese per i prossimi sei anni. Si tratta di un tornante decisivo per il popolo al quale siamo da sempre vicini, che merita finalmente un futuro libero, dopo aver patito innumerevoli sofferenze morali e materiali. Abbiamo sempre ritenuto che l'unica via d'uscita dal grave stato di prostrazione economica in cui versa il Venezuela, dalla profonda crisi sociale che attanaglia la vita dei suoi cittadini e dall'*impasse* politico-istituzionale che il regime di Maduro impone da troppo tempo al Paese, fosse la ricerca di una soluzione pacifica e inclusiva che passasse attraverso un processo elettorale trasparente. Questa Assemblea pochi mesi fa approvò - ci tengo a sottolinearlo - all'unanimità una risoluzione messa a punto della Commissione affari esteri e difesa del Senato, che ho l'onore di presiedere, nella quale si sottolineavano l'urgenza e la necessità di elezioni libere e credibili, oggi, opportunamente, il senatore Casini ha voluto richiamare l'attenzione di questa Assemblea. Va dato peraltro atto al Governo italiano di aver ribadito, in ogni consesso internazionale, l'importanza di non abbandonare il popolo venezuelano dinanzi all'arbitrio del potere, di aver esercitato pressioni per favorire le condizioni minime di riattivazione del libero esercizio dei diritti civili e politici. il percorso che sta conducendo a queste elezioni è stato ed è segnato da violenze, intimidazioni, minacce a tutti gli oppositori e a tutti coloro che sostengono la coalizione che sfida il dittatore Maduro. Anche nelle ultimissime ore, con un'ondata di arresti arbitrari e con una serie di provvedimenti restrittivi, sono stati inferti colpi durissimi, espressamente mirati a diffondere un sentimento di paura tra i cittadini, a frenarne l'entusiasmo e affievolirne la volontà di scrivere una pagina nuova nella storia del Venezuela. Tutto ciò fa seguito all'ingiusta esclusione di Maria Corina Machado, la *leader* più rappresentativa del fronte delle opposizioni, alla quale il regime nei mesi scorsi ha vietato di candidarsi, e a tutti quegli ostacoli con cui si è cercato di rendere difficile, se non impossibile, l'accesso al voto dei venezuelani all'estero, costretti in questi anni ad abbandonare la propria terra per sfuggire a un destino di violenza, di miseria e di sopraffazione. Dei circa 5 milioni di cittadini emigrati, infatti, solo 69.000 sono riusciti a registrarsi per votare e questo la dice lunga sulla natura di un regime dittatoriale che si perpetua in spregio alla volontà popolare, poggiando e anzi alimentando l'incertezza del quadro giuridico, l'inaffidabilità del sistema giudiziario, l'arbitrarietà dell'azione governativa. Ecco perché, soprattutto in queste ore decisive, vanno tenuti bene accesi i riflettori, in modo che a Caracas e in tutti i sobborghi sperduti del Venezuela l'anelito di libertà di quel popolo non perda d'intensità,

dietro ogni progresso ci sono stati l'impegno, il sacrificio, la passione di intere generazioni, di donne e di uomini che non si sono mai lasciati intimidire e che troppo spesso hanno combattuto a mani nude nell'indifferenza generale di altri popoli e di altri Stati, ignari del fatto che ogni limitazione alla libertà, anche nelle aree più lontane, ha ricadute profonde e rappresenta un *vulnus* al grande mosaico della civiltà che tiene unito il quadro globale. Signor Presidente, sono anzitutto grato a lei e ai Capigruppo per l'atto di sensibilità di aver voluto fissare questo dibattito, un giro di opinioni tra i partiti e tra i Gruppi parlamentari sul tema del Venezuela. La collega presidente Craxi ha ricordato la mozione che unanimemente abbiamo approvato nei mesi scorsi. Già nel testo di quell'atto c'è l'auspicio che oggi va rinnovato davanti al Governo.

Consentitemi poi di ricordare a tutti voi i milioni di venezuelani che in questi anni, a causa delle traversie del Paese, sono stati costretti a emigrare in altri Paesi. Pensate a quanti sono in altri Paesi dell'America Latina, che peraltro, con un afflusso così importante di profughi, ha visto destabilizzare la propria economia. Pensate a quanti sono anche in Europa, in particolare in Spagna, e alle migliaia che sono nel nostro Paese. Colleghi, direi che

che si confrontano opinioni diverse. Debbo dire sinceramente che negli anni le opinioni sono sempre meno diverse e sempre più uguali. Ricordo che all'inizio quello del Venezuela era un tema divisivo tra le forze politiche. Oggi è un tema unitivo tra le forze politiche, poiché tutti la pensiamo allo stesso modo. Molti sono palesemente solidali con l'opposizione venezuelana; altri probabilmente avevano delle perplessità in ordine a come l'opposizione venezuelana si stava muovendo; ma tutti, dal primo all'ultimo in quest'Aula,

il potere. Interpretare queste elezioni come una vendetta degli uni sugli altri - argomento che, dal punto di vista emotivo, può anche essere comprensibile - rischierebbe di portare a un arroccamento. Ci deve essere un disarmo. Devo dire che non sempre la giustizia può trionfare a tutto tondo. Probabilmente in certi momenti i compromessi in politica sono inevitabili. Sono belli? No, forse sono brutti. Rispondono alla giustizia e alla moralità al 100 per cento? No, forse non vi vi rispondono. Però pensiamo sempre che di buone intenzioni sono lastricate le vie dell'inferno; per cui se noi, con una rigidità inconcepibile, non dovessimo favorire una sorta di disarmo bilaterale e di passaggio tranquillo di consegne, faremmo soprattutto un grande torto ai cittadini venezuelani. Termino, signor Presidente, citando il Presidente di un grande Paese amico dell'Italia, ma soprattutto vicino del Venezuela, un protagonista della sinistra politica mondiale: Luiz Inácio Lula da Silva. Sapete cosa ha detto nei giorni scorsi? Ha detto una cosa su cui credo possiamo essere d'accordo tutti, davanti ai commenti di Maduro, che diceva sarebbero stati un bagno di sangue e una guerra civile in Venezuela. Ha detto Lula, e voglio terminare con le sue parole, che faccio mie: «Chiunque perda le elezioni deve fare un bagno di realtà, non un bagno di sangue. Maduro deve imparare: quando si vince, si resta; quando si perde, si va via e ci si prepara a disputare un'altra elezione». Lui è esperto, ma credo abbia detto una cosa saggia.

veramente contento di questa occasione e di vedere tutti i colleghi del Senato ricordare le prossime elezioni in Venezuela, elezioni che arrivano da un accordo internazionale che è stato sottoscritto a Barbados e che aveva delle clausole ben precise. Purtroppo quelle clausole sono state violate. Una delle condizioni fissate è che le parti politiche che si sarebbero scontrate in queste elezioni avrebbero potuto liberamente scegliere i propri candidati. Noi sappiamo che le opposizioni saranno rappresentati da González Urrutia, ma González Urrutia non era il candidato delle opposizioni. Maria Corina Machado aveva vinto le primarie con più del 90 per cento dei consensi e il regime di Maduro, con una mossa delle sue, l'ha esclusa dalle elezioni. Machado era stata poi sostituita da Corina Yoris, ma anche Corina Yoris, un'anziana signora rispettabile, amata e tenuta in grande considerazione da tutte le opposizioni, è stata esclusa. Quindi, il candidato che arriva alle elezioni non è né il primo, né il secondo, né il terzo. È un elemento che ci fa ben pensare e ben sperare per queste elezioni? Io direi di no. Ha ragione il presidente Casini a dire che chi perderà dovrà avere l'agibilità di vivere in uno Stato democratico e che non ci siano vendette. Se però il presidente Casini pensava a quello che ci dicono i sondaggi e al fatto che l'opposizione è ampiamente davanti al regime di Maduro, noi purtroppo non possiamo stare tranquilli e pensare che l'esito delle elezioni sarà rispettato, per un semplice motivo: motivo: Maduro non ha mai rispettato la volontà del suo popolo. E lo sappiamo bene, perché Maduro non è nuovo a perdere le elezioni. Ricordiamo quando, per esempio,

al Governo venezuelano: nonostante abbia per esempio cassato la delegazione dell'Unione europea, che si voleva andasse a fare da osservatrice alle elezioni, deve deve sapere che il mondo li sta guardando. Che ci sia o meno una delegazione *in loco*, questo Parlamento e i Parlamenti del mondo libero guardano a quelle elezioni con estrema attenzione, e non soltanto per ragioni politiche, ma anche perché il regime chavista e il regime di Maduro hanno ridotto il Venezuela a carne da cannone. Il Venezuela, da Paese più ricco dell'America Latina, è diventato il più povero. Il Venezuela, grande produttore di petrolio, deve importare la benzina.

continuano le torture, continuano gli arresti illegali, continuano le violazioni. Brogli elettorali si stanno verificando ancor prima che le elezioni si tengano. È stato impedito a quattro milioni di venezuelani residenti all'estero di registrarsi; vengono cambiati i nomi delle scuole, gli indirizzi dei seggi, per fare in modo che i venezuelani non possano andare a votare. a votare. Questo è ciò che io penso. Tutti dobbiamo augurarci che le cose vadano bene; tutti dobbiamo augurarci che, una volta che il regime democratico sia ritornato sia ritornato al potere, un regime veramente democratico, bisognerà assicurare una pacifica transizione, ma giunga un monito da quest'Aula e da tutto il mondo libero al Governo venezuelano: il mondo vi guarda. Sappiamo chi sono i vostri alleati: la Russia, la Cina, l'Iran, gli Stati canaglia, ma io credo che il mondo democratico sia ancora forte abbastanza da far sentire la sua voce e, anche a distanza, anche tenuto fuori da quel Paese, sia in grado di controllare, di verificare e di far sentire la propria voce. Signor Presidente, anche noi siamo molto grati per questo dibattito intorno al 28 luglio e alle elezioni che riguardano il Venezuela. Sappiamo che questa è una stagione nella quale, dalle elezioni negli Stati Uniti, alla guerra in Ucraina, al Medio Oriente, il rischio è di sottacere e di non dare il giusto peso a una scadenza che invece deve rappresentare, come appuntamento veramente democratico, uno spartiacque per il popolo venezuelano fra la dittatura militare di Maduro e l'opportunità che offre la Piattaforma unitaria democratica con la guida di Edmundo González. Purtroppo, le nefandezze di Maduro sono sotto gli occhi di tutti. Dal 2016 guida impunito un Paese, avendo sottoposto nel 2018 i venezuelani a delle elezioni che sono state contraddistinte da brogli e intimidazioni. Il vincitore di quelle elezioni, Guaidó, è stato costretto all'esilio. Sappiamo che Maria Corina Machado e, dopo di lei, Corina Yoris sono state inabilitate e, solo dopo grandi pressioni internazionali, si è giunti alla candidatura di González. Gli Accordi di Barbados non hanno avuto l'effetto sperato. Quindi, perché noi dobbiamo occuparci di un Paese così lontano e di quella data, il 28 luglio? Purtroppo Maduro ha impedito che gli osservatori OSCE e gli osservatori internazionali possano guardare, osservare e vigilare da vicino l'andamento di quell'appuntamento elettorale. Nel frattempo quel Paese è sull'orlo del collasso. Il PIL è caduto dell'80 per cento, come ricordava prima il collega Scalfarotto. La soglia di povertà è intorno al 90 per cento; il salario minimo per i venezuelani è di tre dollari e mezzo al mese.

drammatica di quel Paese. Ovviamente, sono piovute molte condanne internazionali e quello che noi dobbiamo ribadire da quest'Aula è che non lasceremo soli i venezuelani;

Abbiamo trovato persone tutt'altro che rassegnate, persone che credono ancora che l'appuntamento del 28 luglio possa rappresentare un cambio di passo per il Paese. Ecco perché voglio ricordare non contenuti della risoluzione che abbiamo recentemente approvato, ma anche che è nostro compito non solo difendere lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti civili e politici dei venezuelani, ma anche adoperarci affinché i tanti venezuelani residenti in Italia possano esercitare il diritto di voto. E dobbiamo anche tutelare la comunità italiana in Venezuela e le aziende italiane tuttora operanti in quel Paese. Certo, la politica impone anche una dose di realismo e quindi faccio mie le parole e l'auspicio espresso dal presidente Casini: noi non vogliamo una resa dei conti, vogliamo che il Venezuela possa accedere a libere e democratiche elezioni. Non siamo ovviamente ottimisti, ma lavoriamo perché questo possa accadere. Quindi, l'auspicio del presidente Casini è anche il nostro. Noi siamo il Parlamento italiano e oggi vogliamo ribadire che dall'Ucraina al Medio Oriente, passando per Taiwan fino al Venezuela, la difesa della libertà, della democrazia e il rispetto dei diritti umani sono all'apice non solo dei nostri pensieri, ma anche delle nostre azioni. Viva il Venezuela!

che vive attualmente una crisi politica, economica e soprattutto sociale. La popolazione è in fortissima sofferenza e in molti hanno abbandonato il Paese: si parla di 3-5 milioni di persone. Queste elezioni sono importanti. Che siano importanti lo dimostra non solo la nostra attenzione in quest'Aula, ma anche l'attenzione che altri stanno ponendo. Sappiamo che Russia e Cina continuano a sostenere Maduro, vedendo in quel Governo un alleato strategico in America Latina. Mosca ha fornito e continua a fornire supporto sia militare che finanziario, mentre Pechino ha investito pesantemente nel settore energetico venezuelano. In questo scenario, però, va detto che le sanzioni americane pesano moltissimo e sicuramente non hanno aiutato e non aiutano. Mi chiedo se non sia controproducente continuare su questa strada e in realtà se lo chiedono anche gli americani stessi. Ho letto un articolo su «Forbes» di qualche settimana fa che faceva un resoconto della situazione e criticava molto la posizione sanzionista degli Stati Uniti. L'Europa ha sostenuto gli Accordi di Barbados che hanno portato allo svolgimento di queste elezioni, che prevedevano, tra le altre cose - come già accennato dal senatore Scalfarotto - la presenza di osservatori speciali delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e dell'Unione africana. Speravamo che fosse realmente permesso loro di assistere. Sembra però che il Governo abbia ritirato l'invito a tutti gli osservatori speciali. Il clima è surreale: arresti indiscriminati, intimidazioni la dichiarata ineleggibilità della candidata Maria Corina Machado, vincitrice delle primarie delle opposizioni unite, ha obbligato la coalizione a scegliere in poco tempo un diverso candidato - il quarto, come già ricordato la scelta è caduta sul diplomatico, ex ambasciatore, Edmundo González, che da notizie di stampa parrebbe essere in netto vantaggio nei sondaggi. Ricordo che abbiamo avuto l'occasione di confrontarci con la Machado qualche mese fa in videoconferenza. Già allora ci testimoniava la difficile situazione e pochi giorni fa sui *social network* ha denunciato di aver subito un attentato: la manomissione dei freni della sua auto, come se non bastassero gli arresti delle persone del suo *staff* e il mandato di arresto per alcuni deputati. In ultimo, le parole di Maduro durante un evento elettorale a Caracas: un bagno di sangue, se non vincerò, come riportato da RaiNews la settimana scorsa. Parole terribili. Io non sono ottimista, senatore Casini. Mi auguro comunque che venga consentito ai venezuelani di esercitare il diritto al voto, libero e sicuro, anche con riferimento a quei 3-5 milioni di persone che però non potranno farlo. So che alcune organizzazioni internazionali hanno denunciato che la maggior parte di esse verrà esclusa proprio per le regole fittizie e *ad excludendum* imposte dal Governo. Più fonti di stampa riportano ulteriori tentativi del Governo di non facilitare nemmeno le operazioni in Patria del voto. È un eufemismo, per non dire altro.

votate me perché tutti gli altri sotto non esistono. Come ho già detto, non sono molto ottimista. Le premesse non sono proprio delle migliori. Noi possiamo dare un contributo, tenendo alta l'attenzione della comunità internazionale.

all'Assemblea questo importante dibattito. Vorrei esprimere in questa sede tutta la nostra grande preoccupazione e ferma condanna per la grave situazione che sta vivendo il Venezuela, un Paese amico, un Paese amico, che un tempo era prospero e fiorente e che ora è ridotto alla disperazione e alla miseria. Le prossime elezioni rappresentano un momento cruciale non solo per il popolo venezuelano, ma per tutta la comunità internazionale che crede nei valori della democrazia, della giustizia e della libertà. Sotto la dittatura di Nicolás Maduro, il Venezuela è stato trascinato in una spirale di declino senza precedenti. Il regime di Maduro, basato su principi comunisti (sottolineo comunisti) ha sistematicamente violato i diritti umani, represso il dissenso politico e soffocato ogni voce di dissenso e opposizione. Le libertà fondamentali sono state calpestate, la stampa ridotta al silenzio e le istituzioni democratiche erose fino a diventare strumenti nel controllo del potere. I cittadini venezuelani sono stati privati del loro diritto più sacro: il diritto di scegliere liberamente i propri rappresentanti. Le politiche economiche e fallimentari del regime di Maduro hanno portato il Paese alla rovina, paralizzando di fatto l'economia. L'inflazione galoppante ha reso la moneta venezuelana praticamente priva ormai di qualsiasi valore, causando una crisi umanitaria senza precedenti. Milioni di persone sono costrette a lasciare il Paese cercando rifugio in Nazioni vicine e coloro che vi rimangono lottano quotidianamente per sopravvivere tra scarsità di cibo, medicinali e beni di prima necessità. La colpevolezza del regime di Maduro è sotto gli occhi di tutti ed è evidente. Attraverso l'uso della forza, la manipolazione delle elezioni e la corruzione dilagante, ha distrutto le basi della società venezuelana. Il comunismo ha fallito miseramente nel garantire benessere e libertà al popolo venezuelano, portando invece solo oppressione e miseria, come tra l'altro abbiamo visto avvenire in molte altre occasioni storiche. In questa tragica situazione la comunità italiana e quella degli italo-venezuelani hanno sofferto in modo particolare. Migliaia di persone di origine italiana - l'ha detto il presidente Casini che hanno contribuito con il loro lavoro e il loro impegno alla crescita del Venezuela, si trovano ora in condizioni di estrema difficoltà. Le loro attività economiche sono state devastate, le loro famiglie separate e il loro futuro ormai incerto. Molti sono stati costretti a lasciare il Venezuela abbandonando le loro case, i loro affetti, i loro beni, per cercare un rifugio sicuro altrove. Chi è rimasto affronta affronta quotidianamente la mancanza di sicurezza, la scarsità di beni di prima necessità e la continua violazione dei diritti umani. Di fronte a questa drammatica realtà non possiamo rimanere in silenzio. La comunità internazionale deve alzare la voce e fare pressione affinché le elezioni imminenti siano libere, trasparenti e giuste. È imperativo che vengano garantite tutte le condizioni necessarie per un processo elettorale credibile che rispetti la volontà del popolo venezuelano e che permetta il ritorno, come auspicato dai colleghi, alla democrazia. Ho però un grande timore, anzi quasi una certezza, ossia che il regime comunista abbia già agito per negare questi diritti di esercizio della democrazia. Facciamo allora appello agli organismi internazionali, alle organizzazioni per i diritti umani e a tutti i Paesi democratici affinché si uniscano in uno sforzo comune per monitorare le elezioni, denunciare le irregolarità e sostenere il popolo venezuelano nella sua lotta per la libertà. Non possiamo permettere che l'ennesimo atto di prevaricazione passi inosservato. Il Venezuela merita un futuro migliore, un futuro in cui la giustizia e la democrazia prevalgano sull'oppressione e sulla corruzione. È nostro dovere morale sostenere questo cambiamento e lavorare insieme per un mondo in cui ogni essere umano possa vivere in dignità e in libertà. Concludo, Presidente. *Viva Venezuela libre, viva la libertad, abajo el comunismo*. Signor Presidente, ringrazio anch'io i senatori Casini e Craxi per aver voluto questo momento. Credo che sia importante

delle forti ombre. Una cosa certa è che i venezuelani all'estero non potranno votare, benché per la legge venezuelana potrebbero; ci sono già delle forti storture nella fase preelettorale.

l'Assemblea nazionale, poi sciolta da Maduro, aveva eletto come presidente *ad interim* della Repubblica Juan Guaidó, che era presidente dell'Assemblea nazionale stessa. Diversi Paesi europei si erano espressi per riconoscerlo a livello internazionale come il legittimo Presidente *ad interim* in attesa di elezioni regolari, ma la posizione dell'Italia all'epoca impedì all'Unione europea di esprimersi in questo senso. bene che si sappia fin d'ora che l'Italia non sarà indifferente di fronte all'emersione di brogli - che naturalmente auspichiamo non ci siano, ma che di certo quantomeno c'è chi li sta preparando e che saremo conseguenti rispetto a un eventuale verificarsi degli stessi. La dittatura di Maduro, *leader* dal 2008 del Partido Socialista Unido de Venezuela, ha creato danni enormi al Venezuela. Ci sono state addirittura persone morte di fame e migliaia di bambini, privati delle medicine che a loro erano indispensabili, sono morti; milioni di persone sono scappate all'estero: una situazione devastante che colpisce anche i 160.000 registrati con la cittadinanza italiana presso il consolato e il milione e mezzo di e mezzo di venezuelani di origine italiana che sono stimati in quella Repubblica, che avrebbe tutti i presupposti per essere prospera, grazie a un sottosuolo ricchissimo. Una conduzione ideologica fanatica e al guinzaglio di

eque e giuste e, di conseguenza, una ripresa del benessere di quella importante Repubblica.

questo significativo momento di dibattito in vista delle elezioni del 28 luglio prossimo in Venezuela. Devo dire che dobbiamo davvero essere molto orgogliosi di come il Senato della Repubblica, il nostro Parlamento, tenga alta l'attenzione su un Paese così strategico per l'America Latina, così importante per la regione e così pieno di italiani: abbiamo milioni di italo-discendenti in Venezuela e dobbiamo porre la giusta attenzione attenzione per la situazione grave che c'è ed è in atto. Desidero ribadire come il Governo segua con grande attenzione la vicenda venezuelana, anche in ragione degli effetti destabilizzanti della crisi a livello regionale e, come dicevo prima, della numerosissima comunità italiana che lì risiede. Siamo, peraltro, in contatto costante con i nostri *partner* europei e con quelli del G7 per cercare posizioni condivise e per far sentire la nostra voce con sempre maggiore incisività. Anche il ruolo degli attori regionali più vicini al Venezuela, come la Colombia o il Brasile, che, come è noto, detiene la presidenza del G20, è da noi considerato molto importante. Elezioni libere, credibili, trasparenti e competitive, in grado di attivare un processo di riconciliazione politica sono necessarie. È l'unica via attraverso la quale il popolo venezuelano può uscire dall'attuale crisi economica, sociale e umanitaria. Il Paese è entrato nella fase finale (perché mancano davvero pochi giorni) della campagna elettorale e, nonostante il presidente Maduro abbia rispedito al mittente l'invito di una missione di osservazione elettorale dell'Unione europea, come è stato ricordato anche dalla presidente Craxi, l'Italia rimane impegnata in coordinamento con i *partner* per garantire il diritto a un'elezione trasparente, che assicuri il rispetto degli *standard* democratici. È importante che vi siano forme di osservazione elettorale indipendente,

milioni di euro. Infine, come ha sottolineato anche il vice presidente del Consiglio Antonio Tajani, continueremo a vigilare con attenzione affinché da ora e fino al giorno del voto tutte le regole della democrazia siano rispettate. *(Applausi)*.

nel breve periodo di tempo a disposizione, l'8a Commissione è riuscita a svolgere la discussione generale e ad esaminare gli ordini del giorno. Giunti all'esame degli emendamenti, è stato tuttavia inevitabile prendere atto dell'impossibilità di concludere l'esame in sede referente con il conferimento del mandato al relatore. in relazione a quanto riferito dal senatore Rosa, il disegno di legge n. 1197, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44,

pregiudiziale, in quanto abbiamo ravvisato diversi punti di incostituzionalità, a partire dalle premesse. Questo Governo ha presentato questo disegno di legge sulla scorta di tre obiettivi principali: la necessità di dare una risposta certa al crescente fabbisogno abitativo, con il recupero del patrimonio edilizio esistente e la riduzione del consumo di suolo, lo sblocco dello stato di stallo del mercato immobiliare, che risulta penalizzato da incertezze nel quadro normativo di settore che impedisce sia la valorizzazione economica del bene, sia gli interventi di ristrutturazione edilizia. Il terzo obiettivo sarebbe dovuto essere la riduzione del carico degli uffici delle amministrazioni comunali che non riescono a fornire risposte in tempi certi alle richieste di accertamento dello stato legittimo. È stato presentato, questo, come un atto che si limita a sistemare piccole difformità e a regolarizzare questioni meramente formali che creano problemi alla compravendita, al fine per dirla con le parole del Ministro proponente, che ne ha fatto poi solo la cassa di risonanza dello *slogan* lanciato - di risolvere "problemini" di scarsa portata. Tuttavia, il testo che abbiamo ereditato dalla Camera, quindi con le modifiche apportate, reca interventi di ben maggiore impatto, con ricadute sulle variazioni essenziali, sulla doppia conformità e persino sulla parte antisismica della normativa esistente, presentando così un profilo molto più impattante rispetto ad un semplice complesso di piccoli aggiustamenti. Vengono così introdotte misure a regime che si applicheranno senza limitazioni temporali e quindi sprovviste di carattere di eccezionalità e straordinarietà, ponendosi pertanto in contrasto con l'articolo 77 della Costituzione. Il crescente fabbisogno abitativo si dovrebbe affrontare mediante una pianificazione strategica volta all'adeguamento dell'offerta degli alloggi accessibili; anche il dissesto idrogeologico e la sicurezza antisismica nel nostro Paese richiederebbero un intervento urgente, mentre in questo provvedimento non si fa altro che prendere atto del progressivo affermarsi di comportamenti illeciti adeguando la normativa alle condotte illecite e non viceversa. Tra l'altro, è notorio come l'aggravio amministrativo a carico degli uffici comunali sia riconducibile prevalentemente alla grave carenza di personale tecnico nei Comuni e all'esigenza di far fronte alle cicliche sanatorie straordinarie, che hanno nel tempo frammentato e congestionato l'attività delle amministrazioni competenti. Con l'introduzione del silenzio assenso, vengono scavalcate le prerogative di controllo e regolazione proprie delle amministrazioni comunali, andando ad incidere direttamente sul governo del territorio e quindi sulla potestà legislativa concorrente prevista dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione. A titolo di esempio, il superamento della doppia conformità nelle variazioni essenziali consentirà di sanare un aumento consistente della cubatura, modifiche essenziali dei parametri urbanistico-edilizi, ovvero quegli interventi posti in essere in maniera diversa dalla norma assentita, purché risultino conformi solo ed esclusivamente alla normativa urbanistica attuale. In conseguenza di queste scelte i Comuni non potranno neppure condizionare la regolarizzazione dei provvedimenti e degli interventi su opere riguardanti la salubrità, l'igiene, l'efficientamento energetico e l'abbattimento di barriere architettoniche.

per giunta con la diminuzione delle oblazioni. Io non so se vi rendete conto della portata di queste prescrizioni e delle ricadute che le stesse rischiano di avere in termini di sicurezza su tutto il patrimonio edilizio dei privati. Il paradosso è che dopo una norma del genere il Parlamento sarà impegnato a discutere altri vostri decreti che prenderanno in considerazione questioni come eventi alluvionali e dissesto idrogeologico che hanno interessato ultimamente le Regioni. Diciamo che questo è veramente il paradosso. Le disposizioni contenute nel provvedimento risultano altresì in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione sotto il profilo della discriminazione nei confronti dei cittadini rispettosi della legge che non hanno realizzato opere in difformità dalla normativa urbanistico edilizia ed altri cittadini che, al contrario, hanno intrapreso interventi senza il preventivo vaglio degli enti competenti, permettendo loro *ex post* di sanare queste irregolarità. Questa nuova disciplina produrrà, tra l'altro, l'ulteriore effetto di precludere l'applicazione futura di poteri inibitori e sanzionatori previsti a legislazione vigente, con conseguenti ricadute anche sotto il profilo della tutela del territorio, dell'ambiente, della salute e dunque del complessivo assetto dei valori costituzionalmente garantiti ai sensi degli articoli 9 e 32 della Costituzione. Ulteriori profili di illegittimità sono inoltre rinvenibili con riferimento all'articolo 97 della Costituzione e ai connessi principi di ragionevolezza e buon andamento dell'amministrazione. Per la sua scarsa attenzione a livello urbanistico questo decreto-legge porterà una serie di complicazioni interpretative e problematiche applicative che non escluderanno affatto nuovi e maggiori contenziosi. Oltre al contrasto degli articoli della Costituzione già richiamati, le disposizioni contenute nel decreto-legge si pongono in evidente contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità.

ma nel senso di dare la garanzia e la sicurezza ai cittadini che non crolleranno con tutta la casa, con quel solaio o con il soppalco che è stato realizzato abusivamente, che fa volume, incidendo sulla stabilità dell'immobile, per i quali adesso noi diciamo che basta una certificazione per ammetterlo. È davvero una manovra che va ai danni della salute e dell'incolumità dei cittadini. Non serve al fabbisogno abitativo e nemmeno certamente a garantire gli alloggi alle persone.

grandezza dei locali per poterli rendere abitabili, servono a garantire la salute. Quindi abbiamo anche una violazione del diritto di ogni cittadino alla salute, che è un diritto altrettanto garantito dalla Costituzione, uno dei diritti primari. Sbloccare lo stallo del mercato immobiliare? Non lo sblocchiamo certamente così. Lo sblocchiamo con una norma che vuole sanare gli abusi, una norma che ovviamente farà sì che chi li ha compiuti benefici di una sanatoria e chi invece ha rispettato la legge passi come quello che è stato un po' ingenuo a pensare di dover rispettare le prescrizioni. Anche da questo punto di vista ravviso un'ulteriore violazione della Costituzione. Senza contare che la materia edilizia, signor Presidente, è di competenza delle Regioni. Introdurre quindi delle norme così precise e così dettagliate, che vanno a incidere sul testo e quindi vanno a sovrapporsi alla normativa regionale, significa violare la competenza delle Regioni. Il che come sempre - non mancherò mai di farvelo presente, perché francamente mi pare evidente costituisce un modo attraverso il quale si evidenzia la contraddittorietà dell'azione del Governo, tra autonomia differenziata da una parte, che vuole dare autonomia alle Regioni, le quali si trasformerebbero in venti stati in cui ognuno legifera come gli pare (addirittura potrebbero modificare i limiti abitativi e le destinazioni d'uso) e dall'altra uno Stato che ogni tanto ricorre a un decreto d'urgenza (anzi, più spesso che altro) e addirittura pretende di introdurre deroghe alla normativa normativa sull'edilizia. C'è pertanto una violazione dell'articolo 117 della Costituzione e dei principi che regolano la distribuzione delle competenze fra Stato e Regioni. Non ultimo, dire che si introducono queste norme per cercare di alleviare gli enti locali e gli uffici tecnici comunali, che non hanno personale sufficiente per fare gli accertamenti,

così come è palese che dire che non si perseguono gli abusi edilizi e si introduce una sorta di sanatoria *omnibus* perché non ci sono abbastanza impiegati comunali è una violazione dell'articolo 97 della Costituzione e dei principi generali del nostro ordinamento giuridico, che vuole che la legge sia rispettata legge sia rispettata da tutti e che lo Stato garantisca ai cittadini la salute, la giustizia e soprattutto l'efficienza della pubblica amministrazione.

Questo decreto-legge, infatti, è del tutto privo dei requisiti di necessità e di urgenza, posto che contiene modifiche al testo unico dell'edilizia che ben avrebbero potuto essere fatte e apportate con un procedimento legislativo ordinario. Peraltro, si tratta dell'ennesimo decreto-legge sul quale intendete porre la questione di fiducia, secondo una prassi completamente contraria alla Costituzione. L'unica vera e riconoscibile caratteristica di necessità e urgenza riscontrabile in questo decreto-legge è il desiderio, ancora una volta, di produrre un'ulteriore deregolamentazione delle regole edilizie e urbanistiche di governo del territorio, per giunta bypassando l'intesa Stato-Regioni. Proprio voi, che sbandierate con grande forza l'autonomia differenziata, non solo non l'applicate in questo decreto-legge, ma mettete in discussione quella che c'era prima, perché l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione dice che la materia del governo del territorio è attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni. Quindi, non solo voi non rispettate le ulteriori competenze che pure volete regalare alle Regioni, ma neanche quelle che c'erano prima. prima. In sostanza, dite una cosa e ne fate un'altra. Parliamoci chiaro, diciamo chiaramente che, in effetti, questo è l'ennesimo condono, l'ennesima sanatoria spacciata come soluzione che, in

territorio. Invece, sarebbe urgente che un Governo affrontasse finalmente la questione dell'emergenza abitativa, perché ci sono centinaia, migliaia di famiglie che sono senza casa. Ripeto: centinaia, migliaia di famiglie. La metà delle persone che vive in povertà vive anche in povertà abitativa, senza la possibilità di avere accesso alla casa. Contemporaneamente a questo, ci sono 90.000 alloggi alloggi di edilizia economica popolare inutilizzati perché il Governo, ma anche le Regioni in questo caso, non intervengono a fare le necessarie manutenzioni e a completare le stesse abitazioni. Questa è l'emergenza abitativa che bisogna affrontare: come si risana il patrimonio pubblico e come si rilancia l'edilizia popolare per dare risposte alle esigenze di migliaia di famiglie e anche dei giovani, in particolare i giovani studenti fuori sede che cercano casa. Di tutto questo però non si parla. Siamo di fronte al fatto che voi criticate quelli che occupano le case, occupare, in alcuni momenti, è manifestare un disagio che, nella società, è più che giusto: almeno, noi la pensiamo così. Peraltro, ci sono anche

al mercato, al cosiddetto mercato che si regola da solo. Per queste ragioni noi voteremo a favore della pregiudiziale presentata.

dato dalla pioggia di denaro pubblico legato al 110 per cento, oggi ha rallentato e rischia di fermarsi. che cosa vi sia di più urgente di far muovere dallo stallo l'economia del settore dell'edilizia, di far aumentare i posti di lavoro in tale settore. Il decreto, Il decreto, infatti, è stato ribattezzato salva casa per un motivo: perché salva le nostre case da una normativa che, da una parte, è rigida dall'altra, è frammentata, viste le pluralità di competenze divise tra Stato, Regioni e Comuni. In pratica vengono ricondotte a logica, senza precludere le competenze degli enti del territorio, le procedure amministrative incerte che rendono difficili gli interventi sulle case e frenano la commerciabilità dei beni immobili con ripercussioni sui mutui e sulle imposte. Le disposizioni qui previste, che hanno già visto un ampio esame da parte della Camera dei deputati, non contengono condoni palesi, né tantomeno mascherati. Si interviene peraltro solo sulle irregolarità minori e su rigidità normative che hanno messo in difficoltà gli stessi uffici urbanistici comunali, quindi si tratta di semplificazioni necessarie e urgenti. Di tali semplificazioni beneficeranno tutti: gli uffici comunali, i proprietari, gli inquilini che vedono ridotti gli oneri amministrativi, perché ci sarà un mercato più vasto e dinamico sia per le compravendite che per gli affitti. Da ultimo, presentare una pregiudiziale su un decreto-legge che ha avuto un ampissimo accoglimento positivo da parte di tutte le categorie interessate del mondo immobiliare, oltre che dai proprietari e dagli inquilini, che hanno peraltro alla Camera contribuito a migliorare e integrare il testo, significa non capire le esigenze del Paese reale e dei cittadini. Per queste ragioni, noi di Forza Italia, che da sempre siamo i paladini della casa, invitiamo a votare convintamente contro questa pregiudiziale e ad approvare questo provvedimento, che aprirà la strada alla nuova normativa sulla rigenerazione urbana, di cui sono relatore in 8a Commissione, che vedrà città più belle, prestanti, accoglienti e a misura d'uomo.

vanno a regolarizzare difformità dalle variazioni essenziali, tolleranze costruttive ed esecutive, anche legate ai requisiti igienico-sanitari. Tra l'altro, si consente di avere un'agibilità facile per tutti.

misure a regime, applicabili senza limitazioni temporali e dunque sprovviste del carattere di eccezionalità e straordinarietà che consentirebbe di giustificare un intervento normativo sorretto dai presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione. Insomma, questo, assieme a tutto il resto, rappresenta un decreto-legge che contiene un "liberi tutti" inaccettabile, Presidente, anche in considerazione del punto forse più complesso di questo decreto-legge, che è quello relativo al rischio più grande.

Possiamo consentire che, con la conversione di questo decreto, si sancisca il fatto che verrà definito casa uno spazio di 20 metri quadrati?

questione pregiudiziale in esame più che altro perché pensiamo davvero che tra le fila dell'opposizione ci sia un po' di confusione istituzionale

una legge quadro che consente alle Regioni di fare richiesta per avere competenze esclusive in alcune materie che oggi sono considerate concorrenti. Al momento, giustamente, il governo del territorio è una materia concorrente e, stando proprio alla Costituzione, spetta allo Stato

ci può stare, perché quando non si hanno argomenti si ricorre spesso e volentieri a questi artifizi linguistici o a qualche spauracchio, cercando di evidenziare contraddizioni che non ci sono.

non ha alcun fondamento. Infatti, questi decreti vengono convertiti in legge e promulgati dal Capo dello Stato, che è il principale garante del rispetto della Costituzione.

finalmente, ci verrebbe da dire - è un provvedimento a favore dei proprietari di casa dopo le tante penalizzazioni subite

un intervento atteso da migliaia di cittadini - lo sottolineo - che, a causa di piccole difformità interne presenti nella propria abitazione spesso formali e realizzate in anni precedenti, sono sempre rimasti fuori

Sappiamo che si tratta spesso di immobili vecchi, molto vecchi, e soprattutto ubicati nei centri storici. dicevamo, spesso attribuibili all'amministrazione pubblica e anche ad un eccesso di legislazione, perché nel corso degli anni talmente tante sono state le norme e le leggi che

per semplificare - una parola di cui tutti noi politici ci riempiamo la bocca - una volta tanto che arriva un provvedimento che va davvero a semplificare la vita delle amministrazioni pubbliche e di tantissimi cittadini, ci chiediamo come possa essere definito un provvedimento da osteggiare e addirittura che lede il principio costituzionale.

legati alla soprintendenza (e sappiamo le soprintendenze in Italia tante volte quanti meccanismi di burocrazia mettono in campo, che non consentono di spostare nulla). Tutto questo ha bloccato per tantissimi anni

italiana che vede che tutto quello che arriva dall'estero come bello, mentre siamo solo noi quelli brutti che sbagliano, per cui dobbiamo prendere esempio dagli altri Paesi europei. Ebbene, nella stragrande maggioranza dei Paesi europei queste piccole anomalie sono lasciate alla libertà

di questa Europa che tanto sentiamo decantare proprio dagli esponenti che oggi dicono che invece facciamo un provvedimento che non va nella direzione corretta, giusta e di rispetto della Costituzione. Visto che si parlava di enti locali e di Regioni, ricordo che è una norma - perché poi la Lega è un movimento che si mette sempre a difesa e a tutela degli enti locali e delle loro problematiche ed è spesso presente e vicina ai territori - che ha recepito queste lamentele che arrivavano proprio dalle amministrazioni comunali e dalle associazioni che le supportano,

contraddizioni anche delle sentenze dei giudici amministrativi. Addirittura un funzionario comunale si trova nella condizione di ricevere una richiesta di sanatoria di piccoli interventi e di non riuscire a dare una risposta, perché deve districarsi tra una legislazione complicata e giudici amministrativi che intervengono dicendo uno l'esatto contrario dell'altro. non sono solo le sentenze sui balneari che si contraddicono; le sentenze in Italia si contraddicono su tutti gli argomenti (anche questa sarebbe una bella tematica da studiare e quindi risolvere).

alla cerimonia del ventaglio, c'è una contrapposizione sempre più forte: solo perché il provvedimento lo presenta sempre più forte: solo perché il provvedimento lo presenta l'avversario politico, allora non va bene e viene subito demonizzato. la vostra arrabbiatura sia dovuta al fatto che a questo tipo di intervento non ci avete pensato voi quando eravate al Governo.

le due conformità, quella urbanistica e quella edilizia, nel momento in cui viene realizzato intervento rispetto al momento in cui si richiede di sanare l'opera realizzata, anche in

infatti, che i piani urbanistici in questo Paese sono sempre stati espansivi e non regressivi: abbiamo sempre ampliato le cubature disponibili, quindi si può fare un piano in più e, se si è in zona a bassa sismicità, lo si può fare senza nemmeno sottostare alle norme tecniche sulle costruzioni di oggi, quando si costruisce ovviamente agli stati limite ultimi e non alle tensioni ammissibili, come si faceva fino al 2008, quindi senza neanche una verifica che tenga conto dell'azione sismica. anche senza andare in variazione essenziale, ad esempio un piano interrato completo in più, fatto in difformità rispetto al permesso di costruire rilasciato, oggi può essere sanato con il provvedimento in discussione. Io non discuto, possiamo avere posizioni diverse sul

non la vedo come un'emergenza reale del Paese. Tuttavia, a prescindere dal merito e dal fatto che possiamo avere posizioni diverse, almeno vorrei che si dicessero le cose come stanno e che si avesse contezza di ciò che si sta votando. Infatti, sentir dire il presidente

tengo particolarmente non solo per la funzione che svolgo, ma perché avendo fatto il sindaco so bene quanto il tema dei temi che in Italia probabilmente è rimasto sottaciuto per troppo tempo sia proprio quello della sicurezza sismica, in un Paese fortemente sismico, in cui più della metà dei Comuni si trova in una condizione

parte dall'analisi - lo dico rivolgendomi a lei, signor Presidente, ma prendendo spunto da quello che diceva il collega Patuanelli - della questione del rapporto tra sicurezza sismica e sanabilità.

La sanatoria di cui si parla non è un condono, anche se capisco che poi la battaglia delle parole evochi e susciti istinti legittimi nella conflittualità politica, ma le dimensioni del problema sono ben più simili a quelle che il collega Romeo evocava. Cosa succede materialmente quando il signor Mario Rossi si presenta dal responsabile competente del Comune? Posto che le tolleranze sono quelle ricondotte alla modesta entità di cui ripetutamente abbiamo parlato, il tecnico deve prima documentare il fatto che vi sia il rispetto delle norme tecniche vigenti al momento dell'abuso, ma attenzione: è probabilmente sfuggito al collega Patuanelli che proprio dalla valutazione della Commissione competente alla Camera è stato introdotto l'articolo 36-*bis*, che stabilisce che - ed è questo il tema che volevo porre all'attenzione dei colleghi - lo sportello unico, quindi il responsabile tecnico, ove verifichi che esistano problematiche di tipo strutturale, possa imporre e condizionare il rilascio del titolo abitativo all'intervento strutturale che documenti come l'opera

questa procedura a me non è ignota, perché è quella introdotta esattamente nella ricostruzione *post-*sisma del 2016 con un decreto-legge che è stato presentato dal Governo in carica nel maggio del 2018,

che - lo dico apertamente - prima di approfondirlo, anche in me poteva provocare qualche turbamento. C'è un significato politico in questo provvedimento, che ovviamente non è esaustivo di tutte le problematiche che riguardano le rigenerazioni urbane e il rilancio del bene casa. casa. Più volte gli esponenti del Governo hanno chiarito come dovranno essere altri e ulteriori gli elementi da assicurare al *corpus* normativo che regola la casa in Italia per poter arrivare a un risultato compiuto e completo. Questo è però innanzitutto un intervento che va

riuscirà a garantire una maggiore commerciabilità di tutti quei beni sottratti alla possibilità di essere trasferiti o negoziati, specie se afflitti da difformità, e che grazie a questo tipo di intervento potranno essere reimmessi nel mercato, e si tratta di tantissimo patrimonio edilizio. Quale sarà l'effetto, a tutto vantaggio anche e soprattutto delle categorie meno abbienti? Il prezzo del bene casa potrebbe scendere, perché un maggiore inserimento del mercato di beni - questa è una regola troppo elementare anche solo per essere ricordata - può

di un sistema che consente anche di documentare come la salubrità del bene casa possa essere mantenuta e vantata, anche se non completamente ossequiosa di regole del 1975;

proprio con gli avanzamenti delle tecniche costruttive. Dal punto di vista della bioedilizia e dell'utilizzo di materiali innovativi, quante cose sono successe dal 1975 al 2024? Anche da questo punto di vista, quindi, credo che dovremmo ricondurre la valutazione di questo provvedimento a un perimetro più ragionevole. Il bene casa è una scelta politica; per noi la piccola proprietà è un assetto fondamentale della comunità italiana e non abbiamo nessuna paura di iscriversi al partito di coloro i quali considerano la proprietà qualcosa di molto distante non solo dal furto, ma anche da una logica di opportunismo. Vi è poi un secondo tema che non dobbiamo dimenticare. Qui evoco quello che facevo prima di fare fare il senatore, ovvero il sindaco. Ho dovuto combattere contro questa selva oscura di norme che ad oggi regolano la possibilità di sanare e governare le piccole tolleranze. È veramente un viaggio infinito che evoca la possibilità di assunzioni di responsabilità che nascevano automaticamente dal fatto che, nel momento in cui il pavimento normativo è insidioso, sconnesso e incerto, è tanto più grave e probabile che la responsabilità del pubblico amministratore si trovi di fronte a un bivio: non faccio nulla per non rischiare e non firmo oppure faccio, ma avendo sempre negli incubi notturni il rischio di vedermi bussare alla porta per aver introdotto, per una piccola sanatoria per piccole difformità, chissà quale elemento fraudolento nella relazione con il cittadino. C'è anche questo aspetto: semplificare vuol dire ricondurre alla giusta posizione la relazione con i poteri pubblici. Se Se la norma non è chiara e il precetto non è nitido, maggiore è il rischio che il cittadino debba assumere le vesti di suddito rispetto a un decisore politico *(Applausi)* che, qualora volesse

alla soluzione, probabilmente parziale, ma sicuramente necessaria, di una problematica che pochi conoscono

ha già pagato e, ove la sua pratica fosse respinta, dovrebbe reclamare denaro e risorse ripetute dall'erario comunale. Questo è un problema che, con ogni probabilità, cuba più di un miliardo,

decine e decine di migliaia di case che non sanno se vivono in un regime di regolarità urbanistica ed edilizia o meno. Sembra una cosa assurda, ma in parte questo provvedimento si riferisce al patrimonio di decenni fa; non parliamo del nuovo, della configurazione edilizia e della rigenerazione urbana, ma di come mettere mano a un grande problema, che determina l'impoverimento dei legittimi proprietari di una casa e che fa salvo comunque e sempre il principio della sicurezza sismica e che quindi va annoverato a buon diritto fra l'insieme dei provvedimenti che ispirano questo Governo, che fa della semplificazione e della tutela del cittadino e della proprietà uno degli elementi cardine della sua proposta politica. È su queste premesse che, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia, dichiaro la totale e convinta contrarietà alla questione pregiudiziale proposta.

Com'è emerso anche dal dibattito appena terminato sulla questione pregiudiziale, la maggioranza continua ad andare avanti a testa bassa e anche questo provvedimento, sul quale…

Com'è emerso anche ieri nella Conferenza dei Capigruppo, il Partito Democratico, così come tutti gli altri Gruppi di opposizione, aveva chiesto un confronto in quest'Aula con il vice presidente e ministro delle infrastrutture Salvini, che però evidentemente non avverrà nemmeno oggi, perché il Governo ha scelto di porre la questione di fiducia, signor Presidente, sulla maggioranza stessa. Mentre facevamo questo dibattito, signor

che definisce il grado di civiltà di un Paese o almeno di civilizzazione di una società, che si misura anche dalle carceri (purtroppo, il nostro grado è molto basso). Signor Presidente,

la Commissione giustizia ha abdicato alla sua funzione, le chiediamo di accelerare l'arrivo di questo provvedimento in Aula e di far venire il ministro Nordio in Aula, visto che non abbiamo il piacere di confrontarci con lui e, men che meno, con le strutture. Abbiamo saputo infatti che questa mattina la presidente Bongiorno si è confrontata addirittura con il ministro Nordio e con il sottosegretario Delmastro,

che non può essere sottaciuto e che non può passare in una logica di archiviazione rapida. Signor Presidente, eravamo entrati in questo dibattito

andavano nella direzione di recepire un disegno di legge presentato alla Camera dal nostro collega Giachetti sulla riduzione dei termini per la liberazione anticipata. Ora sta accadendo una doppia operazione alla Camera, si vuole rimandare in Commissione il disegno di legge Giachetti per impedire che possano essere espressi voti segreti, voti segreti, che farebbero emergere una divisione all'interno della maggioranza; qui, si sbatte la porta in faccia rispetto a una discussione di merito,

l'opposizione e vi siete chiusi a riccio per tentare di riuscire a trovare un punto di coagulo tra le due anime della maggioranza. Il risultato è che arriva un decreto-legge monco e annacquato, che non risolverà in alcun modo il problema drammatico delle carceri e soprattutto che impedisce a quest'Assemblea di esprimersi su questioni di merito. Pertanto, signor Presidente, nell'associarmi alla proposta del presidente Boccia,

dicevo, riteniamo indispensabile che la discussione in ordine al decreto carceri sia la priorità dei nostri lavori.

la capacità di risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri, per poi scoprire che quella collaborazione richiesta in Aula veniva in qualche modo depredata di ogni contenuto in Commissione, quando il

sconveniente per il rispetto istituzionale che ci dev'essere tra colleghi, in particolare della Presidenza della Commissione - scopriamo dalle agenzie che il tema politico che divideva ancora una volta la maggioranza rispetto agli emendamenti presentati da Forza Italia è stato risolto con alcune riformulazioni, quindi «tutto va bene, madama la Marchesa». Ecco, forse

Visto che dite continuamente di essere un Governo politico e di avere una maggioranza, fatela valere, ma non sempre con decreti imposti con la fiducia.

luogo, con riferimento all'intervento del senatore Patuanelli, è stato detto che non c'è stata correttezza istituzionale, perché sono state annunciate alle agenzie alcune riformulazioni che era il caso di annunciare in Commissione. Errore:

secondo luogo, con i giornalisti si è parlato dopo l'approvazione di queste riformulazioni. Passiamo alla correttezza dei lavori in Commissione: c'è stato un ampio dibattito (ore ed ore di dibattito) e i relatori hanno garantito ascolto; dopodiché, una serie delle proposte che erano state fatte, che sono condivisibili, secondo me, dall'intero arco costituzionale, sono in realtà state inserite dal Governo negli emendamenti che sono stati presentati lunedì, quindi l'ascolto c'è stato e poi il Governo ha preso atto delle proposte avanzate infine, su altri emendamenti ci sono stati ascolto, ma non condivisione, e ampio dibattito. Allora, se per regolarità dei lavori intendiamo che necessariamente i relatori devono accogliere alcuni emendamenti, la risposta è che non c'è stata condivisione e non sono stati accolti. Ma, siccome per me correttezza dei lavori significa dare la parola, ascoltare e cercare di migliorare un testo, e poi essere liberi anche di dire no,

rendiamo un grande servizio agli italiani. Si tratta davvero di un provvedimento salva casa degli italiani. Le premesse per sostenere questo provvedimento sono presto dette.

Circa 6 milioni di case italiane sono state costruite prima dell'entrata in vigore della legge Bucalossi del 1977 e prima del decreto ministeriale sanità del 5 luglio 1975 sulle altezze minime e sui requisiti igienico-sanitari. Quasi cinquant'anni sono passati, il mondo è cambiato e non possiamo far finta di nulla. A questo stato di fatto del nostro patrimonio immobiliare dobbiamo aggiungere le difficoltà di reperimento delle pratiche edilizie negli archivi comunali e la mancata autorizzazione delle varianti in corso d'opera, che non era contemplata nella normativa ante 1977. Nel recente passato abbiamo chiesto agli italiani di svecchiare le loro case, ammodernarle, efficientarle e renderle antisismiche. Se da un lato abbiamo chiesto agli italiani di spendere i soldi per rendere più efficienti dal punto di vista energetico le loro case, per tutelare l'ambiente e non consumare ulteriormente il suolo - è una risorsa finita - dall'altro lato, non lo abbiamo consentito loro, perché quelle stesse abitazioni che chiediamo di recuperare non sono conformi a normative che spesso non erano neanche in vigore quando sono stati costruiti gli immobili. Quindi, questo provvedimento davvero non fa altro che salvare milioni di case degli italiani, consentendo di superare piccole difformità. Stiamo parlando non di abitazioni costruite senza titolo edilizio - dobbiamo ricordarlo - ma di abitazioni costruite legittimamente e che, per i più svariati motivi, presentano delle piccole difformità. un esempio per tutti. Pensiamo a una famiglia che acquista una casa, magari con grandi sacrifici, composta da due camere da letto, una per i genitori e una per il figlio. Quando nasce il secondo figlio cosa fa? Acquista una nuova casa? possibile se ha la disponibilità, ma di sovente fa costruire una parete di cartongesso e crea una nuova cameretta. Ritengo che tutti coloro che in quest'Aula hanno onestà intellettuale converranno sul fatto che non si tratta di un abuso edilizio equiparabile, ad esempio, alla costruzione di una villa con piscina sulla spiaggia. Stiamo parlando di una piccola modifica, che però rende l'abitazione difforme dal titolo edilizio e che comporta una serie di problemi al cittadino perché ne impedisce la vendita, l'affitto o anche la possibilità di efficientarla dal punto di vista energetico. Pensiamo anche agli immobili ereditati dai nonni e costruiti in un periodo in cui la preoccupazione era avere una casa e non una casa che fosse perfettamente in regola. Non dobbiamo dimenticare, poi, che queste piccole difformità problemi non solo al cittadino, ma anche ai nostri Comuni che sono intasati di pratiche che non vanno avanti. Con questo provvedimento quindi, da un lato, sgraviamo gli uffici comunali di tutta una serie di pratiche ferme da anni; dall'altro lato, mettiamo in condizioni il cittadino non solo di godere appieno del proprio immobile, ma anche di poterne disporre liberando migliaia di immobili, che magari sono vuoti perché non possono essere venduti per lievi difformità, e immettendoli sul mercato. Questo significa ridurre il consumo del suolo, perché parliamo di immobili che già esistono e che spesso sono ubicati nei nostri centri storici; centri che si vanno svuotando sempre di più, anche perché il patrimonio immobiliare è fermo per questioni di conformità edilizia. È chiaro che si tratta - è bene ripeterlo - non di dare il via libera ad abusi di tutti i tipi, ma di consentire l'uso di immobili esistenti che sono legittimamente costruiti e sono lievemente difformi al titolo edilizio. È altrettanto chiaro che si tratta non di una riforma strutturale, di cui pure ci sarebbe bisogno visto che il testo unico risale a ventitré anni fa, ma di una misura urgente per risolvere situazioni diventate intollerabili in uno Stato civile. È utile evidenziare come l'8a Commissione sia già impegnata per arrivare a definire un provvedimento che tratta del tema della rigenerazione urbana, a conferma che certi temi vanno affrontati. Il Governo Meloni, come i cittadini italiani stanno apprezzando da due anni a questa parte, è il Governo delle azioni concrete, che assume le decisioni e lo fa ascoltando tutte le parti coinvolte, agendo in modo deciso e rapido. È il Governo che oggi vuole rimuovere quei piccoli ostacoli che impediscono al cittadino di godere del proprio immobile. Abbiamo ascoltato le critiche dell'opposizione e la sua solita demagogia ideologica del no a prescindere ai provvedimenti del Governo. Devo dire che ancora una volta non si smentisce e continua ad avere posizioni del tutto disancorate dalla realtà e lontane anni luce dalle esigenze dei cittadini. Non avete ancora imparato. Negate la necessità di questo provvedimento e mentite agli italiani facendo finta che il problema non esiste. Dite chiaramente agli italiani da quale parte vi ponete: risolvere i problemi o dire no a prescindere perché siete opposizione? L'Italia non può rimanere ferma a decenni fa perché nessuno ha avuto il coraggio di prendere in mano le situazioni e risolverle. Questo è, quindi, un provvedimento concreto che va incontro alle esigenze degli italiani, che semplifica la vita degli italiani, che crea una reale possibilità di crescita per gli italiani e per il nostro Paese.

culturalmente è una rivoluzione liberale: ecco come il ministro Salvini ha definito il provvedimento in esame, che ha fortemente voluto per andare verso la semplificazione, agevolando amministrazioni e cittadini. Parlare di edilizia e di immobili esistenti significa parlare La burocrazia sta uccidendo il Paese: i nostri uffici comunali vivono sommersi di pratiche che non riescono a trattare e i cittadini sono costretti ad aspettare da anni risposte che faticano ad arrivare. La politica della Lega è stata sempre per la gente, è una politica di territorio, non per sanare certamente tutti gli abusi, come dicono i detrattori di questo provvedimento. Forse siamo in ritardo, sì, forse l'Italia è in ritardo; evidentemente ci voleva Salvini per arrivare a fare quello che in tanti Paesi europei è già realtà. È un intervento che entrerà nelle case di milioni di italiani in maniera positiva e risolutiva. Per la pubblica amministrazione, passiamo dal silenzio rigetto al silenzio assenso. Si liberano i Comuni da valanghe di pratiche stimate in 4 milioni: il Comune incassa, il cittadino paga e rientra in possesso del suo bene. Allo scopo di offrire una soluzione alle numerose esigenze rappresentate dagli attori coinvolti il presente decreto-legge reca disposizioni di carattere urgente volte a fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo, supportando però al contempo gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo. In particolare, le nuove misure sono finalizzate a rimuovere quegli ostacoli ricorrenti nella prassi che determinano lo stallo delle compravendite, a causa di irregolarità soprattutto formali. Si tratta di misure finalizzate, quindi, a tutelare i proprietari che, avendo legittimamente acquistato immobili in assenza di irregolarità risultanti da atti pubblici, si trovano oggi nell'impossibilità di alienare i propri immobili in forza delle normative sopravvenute. Questo anche nell'ottica di stimolare un andamento positivo dei valori sia di acquisto che di locazione dei beni immobiliari residenziali. decreto-legge trovano le proprie ragioni di straordinaria necessità e urgenza nell'esigenza di sbloccare situazioni di totale stallo in cui oggi versa il mercato immobiliare, fortemente penalizzato dalle incertezze del quadro normativo di settore, che difficilmente consente di dimostrare lo stato legittimo di un immobile, inibendo la valorizzazione economica del bene e anche la possibilità di interventi di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico.

Questa volta l'intervento del Governo in materia edilizia era tanto atteso da migliaia di cittadini che, a causa di piccole difformità presenti nella propria casa, sono rimasti sempre fuori dal mercato immobiliare o da incentivi e *bonus* edilizi. L'intervento del Governo, in particolare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, era tanto atteso e opportuno anche ai fini del conseguimento degli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo. Infatti, della necessità di limitare il consumo di nuovo suolo agricolo e di costruire nell'edificato si parla sempre da tanto tempo, ma la mancanza di norme appropriate per la demolizione e la ricostruzione degli immobili ne ha spesso bloccato la realizzazione. Negli ultimi anni le amministrazioni comunali - e qui andrebbe fatto veramente un applauso ai tanti coraggiosi sindaci che sono tutti i giorni in trincea si sono dovute districare con le contraddizioni delle sentenze dei giudici amministrativi per risolvere la complessità delle casistiche che si presentano su edifici sia privati che della della pubblica amministrazione. Spesso si sono verificate situazioni in cui le amministrazioni comunali hanno evitato di intervenire su immobili che non potrebbero regolarizzare, lasciando indenni interventi attualmente illegittimi nelle periferie delle città, perché magari hanno ritenuto illogico ordinare la demolizione per difformità presenti nell'edificio rispetto alla disciplina urbanistica e edilizia vigente al momento della realizzazione dello stesso, per poi consentirne la ricostruzione identica in quanto conforme alla normativa urbanistica vigente. Il decreto-legge in esame agevola la realizzazione di investimenti e la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, sostiene la ripresa economica e produttiva e attua uno snellimento - questa è la cosa che più ci interessa - e un'accelerazione dei provvedimenti amministrativi in materia urbanistica e edilizia, riducendo oneri e adempimenti. In conclusione, come dicevo prima, il testo unico in materia di edilizia del 2001, vecchio ormai di più di vent'anni e più volte modificato da decreti-legge negli ultimi anni su più parti, manca di concretezza e di risposte immediate alle necessità del nostro patrimonio edilizio. Del resto, si tratta di un decreto del Presidente della Repubblica che ha cercato di convogliare in un testo unico disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, tenendo conto della frammentazione legislativa degli anni precedenti, dove un gran numero di Comuni non era provvisto di piani regolatori generali approvati e spesso neanche di piani di D'altra parte, l'evoluzione tecnologica negli ultimi anni ha fatto emergere imprecisioni sulle misure degli edifici realizzati negli anni passati nell'altezza, nei distacchi, nella cubatura, nella superficie coperta, che, quando vengono valutati rispetto a una superficie di modesta entità spesso, impattano per più del 2 per cento del totale consentito dalle norme del testo unificato e bloccano qualsiasi commercializzazione dell'immobile. Basta ricordare tutte le difficoltà che hanno trovato i cittadini nell'usufruire delle detrazioni fiscali del 110 per cento, dove la possibilità di intervento si è scontrata con una serie di difformità edilizie nelle costruzioni che, nonostante potrebbero essere risolte proprio utilizzando le possibilità previste dall'articolo 36 del testo unico dell'edilizia, non hanno potuto esserlo per le difficoltà connesse alla norma. Infatti, Governo e Parlamento sono intervenuti con modificazioni della legge del 2020, assoggettando a comunicazione di inizio lavori avvenuta (CILA) gli interventi del superbonus, anche qualora abbiano riguardato le parti strutturali degli edifici o i prospetti, superando l'obbligo della doppia conformità edilizia e l'attestazione dello stato legittimo dell'immobile e annullando la decadenza del beneficio fiscale in caso di difformità. In pratica, sono rimasti esclusi dal beneficio gli abusi totali sprovvisti del titolo abilitativo originario o di quello che ha sanato l'assenza di un titolo abilitativo originario, mentre sono stati ammessi al superbonus tutti quegli immobili che presentano difformità parziali grandi o piccole. Per tutte queste ragioni e per altre ragioni che sono contenute negli emendamenti che i nostri colleghi del Gruppo Lega-Salvini Premier hanno introdotto in Commissione ambiente alla Camera, il nostro Gruppo è fermamente favorevole alla conversione in legge del presente decreto.

ritengo che il riferimento ai sindaci sia assolutamente pertinente: anch'io ho fatto il sindaco e so che cosa vuol dire affrontare situazioni in cui la complessità delle norme rende assolutamente difficile, quando non impossibile, risolvere i problemi del cittadino. qualche riflessione sulla proprietà edilizia privata nel nostro Paese credo che sia necessario farla. Lungi da me volere dei proprietari di casa italiani che sono - lo ricordo - oltre il 70 per cento del totale, quando in altri Paesi d'Europa sono molti di meno: in Germania il 45 per cento, in Danimarca addirittura meno del 40. Non è che sia un merito o un demerito essere padroni della propria casa, ma è un'abitudine che porta a delle conseguenze, le

per cento del totale delle case che si trovano oggi in Italia e vengono costruite, ovviamente, all'inizio investendoci tanto e poi "sparagnando", tant'è che negli ultimi decenni del Novecento sono state fatte grandi quantità di case ed edifici che sarebbero già

che dobbiamo spendere soldi per comprare la casa, ma non ci poniamo il problema dei soldi che spenderemo poi per mantenerla. Quando uno compra un'automobile, sa che, se ne compra una molto costosa, spenderà poi tanti soldi anche per mantenerla. Invece, quando uno compra la casa, a prescindere

tanti proprietari oggi in Italia che posseggono e abitano case che sono qualitativamente scadenti; ciò vuol dire che spendono un sacco di soldi per energia, energia, riscaldamento e raffrescamento. E sono spese maggiori di quelle che sostengono altri proprietari in altri Paesi d'Europa più attenti alla qualità dell'edilizia. dovrebbero fare degli investimenti per migliorare la qualità di quelle case, ma non hanno i soldi per farlo. Questo è il vero problema del nostro Paese. È un problema che nessuno analizza. Se andate a guardare le statistiche del Censis Censis o altre autorevoli ricerche che vengono condotte sul patrimonio edilizio, non si trova traccia di analisi di questo tipo. Non è mica bello andare a mettere il naso sulle questioni, è bello poter dire che i proprietari di casa fanno un investimento per la vita. È bello, ma non è quello che serve per far stare meglio gli abitanti del nostro Paese. Questo è il vero problema che non viene risolto con la norma in esame.

Ciò però non deve far dimenticare che ci sono anche persone che costruiscono rispettando le regole e che ogni volta che c'è una sanatoria noi aiutiamo, invece, anche quelli che le regole non hanno rispettato. Ma soprattutto non ci poniamo il problema di evitare la prossima sanatoria. Andando avanti così, fra vent'anni avremo un'altra sanatoria perché non abbiamo fatto nulla per evitare che si perpetui nel tempo l'errore che hanno commesso quelli che c'erano prima di noi. Questo secondo me è assolutamente folle. Dovremmo invece ragionare seriamente su come mettere mano al patrimonio edilizio italiano, che ripeto che è scadente. Oltre l'80 per cento delle case non supererebbe le soglie di qualità minime per ottenere i certificati che da noi si chiamano casa clima e altrove si chiamano in altro modo, ma sono comunque certificati di qualità. Questo provvedimento non fa nulla in questa direzione. Questo è quello che manca. La politica - secondo me - deve guardare lontano. Noi non stiamo guardando lontano: stiamo guardando vicinissimo, anzi, stiamo guardando negli uffici dei Comuni per toglierci il problema delle carte accumulate. È importante, ma non è tutto. Sono convinto che bisognerebbe fare un salto di qualità e questa discussione, e in particolare il fatto che si vada verso una fiducia, non lo farà fare e mi dispiace molto.

provvedimento che oggi stiamo esaminando rappresenta sicuramente un grande intervento che produce all'interno del testo unico dell'edilizia importanti Ho ascoltato il dibattito sia in Commissione sia quest'oggi alla Camera e ho trovato pesanti osservazioni da parte delle opposizioni su questo decreto-legge, che addirittura ci accusano di inserire dei condoni edilizi. Sono tutte accuse che meritano necessariamente una smentita e una risposta, perché evidentemente i rappresentanti del centrosinistra non hanno capito

proprietari di immobili che noi intendiamo tutelare anche rispetto a quello che è un tema molto caro ad alcuni rappresentanti del centrosinistra. Mi riferisco alle occupazioni abusive. E allora occuparsi della regolarizzazione e delle lievi difformità edilizie vuol dire riconsegnare al mercato immobiliare molti immobili, consentire loro la ristrutturazione e, nel tempo della transizione verde, consentire anche lavori di efficientamento energetico. Questo provvedimento, dunque, introduce tutta una serie di misure fondamentali, che erano attese dai cittadini da anni. Soprattutto, questo provvedimento crea le necessarie condizioni per mettere a disposizione degli italiani uno straordinario patrimonio edilizio esistente, ad oggi non utilizzato o scarsamente utilizzato. Parliamo di unità abitative e di immobili che si renderanno immediatamente disponibili su tutto il Paese, in sintonia con quello che è il tema di oggi, ovvero la riduzione del consumo del suolo. Non si tratta quindi di alcun condono edilizio. Il decreto salva casa, con le sue semplificazioni, con la modifica delle tolleranze di costruzione e agevolando i cambi di destinazione d'uso, libera immobili sul mercato, regolarizzandoli, permettendone la vendita o accelerandone il necessario processo di riqualificazione, interrotto, ad esempio, per mancanza della doppia conformità. Sono tutti aspetti che dovremmo conoscere bene, perché ce ne siamo già occupati per agevolare e sbloccare i processi di ricostruzione dovuti alle varie calamità che hanno colpito la Nazione, e lo ricordava prima il commissario Castelli. Con il decreto oggi in discussione viene superato il vecchio istituto della doppia conformità, limitatamente ad alcuni casi. La vecchia formulazione dell'articolo 36 del testo unico dell'edilizia infatti, che disciplina l'accertamento di conformità - lo strumento tipico per sanare le difformità edilizie - è stato nella realtà, fin dall'inizio, di difficile applicabilità. Di conseguenza ci sono molti manufatti, in genere costruiti vari decenni fa, che sono in una sorta di limbo, perché sono formalmente regolari, non sono suscettibili di interventi di riqualificazione e, quindi, non sono commerciabili. In relazione a questi le amministrazioni comunali non possono assumere alcuna iniziativa sanzionatoria, perché sul piano amministrativo non c'è conoscenza del loro stato.

Ricordo a me stesso che i partiti delle opposizioni, che oggi gridano allo scandalo, si sono anche loro cimentati, quando erano al Governo, con la revisione delle tolleranze edilizie, ampliandone la portata. Parlo del decreto semplificazioni del 2020, fatto dal Governo Conte II; in maggioranza c'erano il MoVimento 5 Stelle, il PD e Italia Viva. Se ne sono occupati perché, nell'applicazione del famigerato

conformità del nostro patrimonio edilizio, che di fatto non rendeva applicabile il provvedimento di cui ancora oggi stiamo contando i danni. Lo stesso discorso vale per il recupero abitativo dei sottotetti, che qualcuno magari può considerare come un condono, ma che invece viene inserito all'interno del provvedimento per cercare di risolvere il dibattito che c'è su questo tema

stanno legiferando in maniera autonoma. Ai partiti delle opposizioni, che oggi accusano di sanare i sottotetti, ricordiamo che in molte Regioni esistono leggi che vanno in questa direzione, introdotte proprio da Governi di centrosinistra. È il caso dell'Emilia Romagna, che ha una legge sul recupero dei sottotetti dal 1998 (ovviamente governava il centrosinistra); oppure della Campania, nel 2000 (anche lì c'era un Governo di centrosinistra), o della Basilicata, nel 2002 (anche qui con una maggioranza di centrosinistra), e così via. In Puglia, nel 2007, governava il centrosinistra; nel Lazio c'è una legge analoga dal 2009, e anche in questo caso con un Governo di centrosinistra; nella rossa Toscana, con una legge del 2010; nelle Marche, con il centrosinistra troviamo una legge sui sottotetti dal 2015. In Umbria esiste una legge dal 2015 sui sottotetti, e anche in questo caso con un'amministrazione di centrosinistra, e così via: in Sicilia dal 2016, in Piemonte dal 2018, tutte con Governi di centrosinistra. *(Applausi)*. Regioni che hanno una legge sui sottotetti, ben dieci sono state attivate da amministrazioni di centrosinistra. Dunque, se dovessimo credere alla tesi delle opposizioni, che il recupero dei sottotetti equivale a un condono, potremmo dire, senza paura di essere smentiti, che sono proprio i partiti di centrosinistra a sponsorizzare i condoni edilizi nelle Regioni italiane. *(Applausi)*. Sappiamo, invece, che questi provvedimenti sono sono destinati a cercare di colmare un fabbisogno abitativo. Così come non rappresenta una sanatoria edilizia l'ampliamento delle categorie di di interventi di edilizia libera, ovvero tutte quelle categorie di interventi edilizi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abitativo: estendere anche ai porticati la possibilità di realizzare, in aggiunta ai balconi, le cosiddette Vepa, vetrate amovibili e totalmente trasparenti; oppure realizzare

data ai tecnici abilitati, di asseverare l'agibilità per locali con altezza di 2,40 metri e di alloggi monostanza di superficie di 20 per una persona e 28 metri quadrati per due persone. Chi conosce il patrimonio edilizio italiano sa perfettamente che, nel tempo, ha subito delle lievi modifiche interne ed esterne, realizzate non da feroci speculatori edili, bensì da padri di famiglia, per cercare di adattare il proprio appartamento alle mutate esigenze familiari, magari per realizzare una camera da letto in più per il proprio figlio, per ampliare una finestra per garantire maggiore luminosità. È a queste persone che si rivolge il decreto, per cercare di sanare piccole difformità edilizie, andando ad ampliare le tolleranze, così come è stato fatto anche dal centrosinistra dal centrosinistra in passato. Signor Presidente, è un provvedimento assolutamente sociale questo voluto dal Governo Meloni. È un provvedimento utile, perché interviene sull'esigenza abitativa di tantissimi italiani. È necessario, perché semplifica la normativa alleggerendo anche il lavoro degli uffici tecnici, dando certezza economica e valore al patrimonio esistente. È un provvedimento che non prevede oneri aggiuntivi allo Stato, bensì nuove entrate, soprattutto per i Comuni, e che destina parte di esse a interventi a interventi di natura ambientale come l'abbattimento di abusi presenti sul territorio comunale e opere di rigenerazione urbana. Soprattutto, è un provvedimento che dà la possibilità alle nostre unità abitative, alle nostre case, al nostro patrimonio edilizio di poter usufruire di tutta una serie di interventi edilizi per andare

la casa nasce con l'uomo, anzi l'uomo, la persona, nasce quando sceglie di lasciare

Noi ce ne intendiamo molto di case sia dal punto di vista della creazione di abitazioni, sia per la bellezza della casa, qualsiasi casa.

rappresenta intanto una garanzia psicologica di serenità maggiore. Non ci si sente più nemici degli altri, del condominio, del quartiere, tra parenti. Permette di liberare il mercato e, quindi, di abbassare - paradossalmente, ma non tanto - il prezzo delle case, diminuire l'abusivismo e garantire maggiore serenità. Come si fa a dire no ad un provvedimento che permette anche di rigenerare un rapporto, spesso complesso, tra amministrazioni locali e cittadini? Siamo tutti un po' folli. Io faccio lo psichiatra nella vita e rispetto la follia, ma magari in quest'Aula cerchiamo di non usarne troppa. Insisto nel dire che permettere la normalizzazione di piccole difformità è un atto liberatorio e civile. Dire di no è come dire di no a una maggiore pace con sé stessi, con la famiglia, con l'ambiente di vita. Davvero non riesco a comprendere. Come ha Come ha detto il collega che mi ha preceduto, tutto il discorso della sanatoria dei sottotetti è voluto soprattutto dalla sinistra

lasciamo perdere queste battute - non può esistere una doppia verità. Se il centrosinistra fa una cosa, è buona; se la fa il centrodestra, è una schifezza. Ragazzi, capisco un po' di variabile - come dire - partitica, ma essere totalmente contrari ad una cosa facile da comprendere, oppure dire sì solo se lo facciamo noi, a me sembra un po' una ciofeca della politica. Vorrei terminare dicendo una cosa, Presidente, e la dica anche ai colleghi. Esistono centinaia di migliaia di cittadini che, vuoi per mancanza di mezzi economici, vuoi per mancanza di informazioni, avendo una disabilità in casa… si dice, eccolo quello, parla sempre di disabilità, ma no, io considero razzista l'obbligo che una persona con disabilità parli solo di disabilità … mi verrebbe l'ansia, la claustrofobia psicologica, però quando ci vuole ci vuole, Presidente. Tanti genitori di persone con disabilità che non usano i moderni strumenti di abbattimento delle barriere architettoniche, come non si usano strumenti moderni anche per le piccole abitazioni, nel fai da te commettono qualche piccola infrazione che però permette la libertà del cittadino con disabilità. Uno scivolo in più, l'abbattimento o l'allargamento di una porta, provocano libertà.

forse perché mi sento bugiardo, o forse perché faccio il neuropsichiatra - che aveva fatto un bellissimo scivolo di legno per permettere anche alle persone con disabilità e agli anziani di entrare in questa meraviglia,

ha permesso a sé stesso o ha ereditato piccole difformità e per questo vive nell'angoscia o nell'impossibilità di vendere, di creare un mercato, perché compiremmo un'azione ingiusta, immotivata e veramente

che ha troppe scosse telluriche non solo fisiche, ma anche psicologiche. Vorrei terminare anch'io ricordando il Venezuela, dove andai per la prima volta quasi mezzo secolo fa e dove sono stato accolto benissimo da tanti venezuelani e da tanti italiani. Riuscii, perché camminavo abbastanza bene, ad andare anche in Amazzonia. In quel periodo scoprii i *murales* che in Italia non conoscevo del tutto, magari conoscevo C'era un termine che mi ha affascinato da sempre in quel Paese meraviglioso che è anche in parte nostro: *adelante pueblo*, per manifestare la voglia di libertà. Vorrei che anche noi ci unissimo, come abbiamo fatto in maniera esemplare e corale stamattina, alla voglia di libertà di questo meraviglioso Paese. *Adelante pueblo!* Lo possiamo fare anche dicendo bugie, a livello di questo decreto-legge

e quello della proprietà immobiliare e degli inquilini. Cominciamo con l'edilizia. In questi anni l'edilizia ha dovuto trasformarsi, perché sul fatto che non dobbiamo più consumare nuovo suolo penso che siamo tutti d'accordo. È evidente che l'edilizia ha reagito a questo trasformandosi. C'è che si è specializzato nei lavori pubblici e c'è chi si è specializzato in ristrutturazioni. Questo settore è stato illuso, soprattutto nel periodo del superbonus al 110 per cento, quando c'è stata un'iniezione enorme di denaro pubblico sostanzialmente per efficientare le case, ma che comunque rientrava in quella che è la ristrutturazione edilizia. È un settore che adesso è in crisi e in difficoltà, rischia di perdere non solo aziende, ma decine di migliaia di posti di lavoro. salva casa aiuta sicuramente in parte l'edilizia ad avere nuovo stimolo e nuovo lavoro, ovviamente se questo decreto-legge viene inteso come il primo passo, quello urgente, per iniziare a ripensare le nostre città. Qui mi collego con riforme più ampie, come quella della rigenerazione urbana di cui stiamo parlando in 8a Commissione. Il fatto che ci siano otto disegni di legge

In Italia il proprietario è una figura vessata, non solo dalle tasse che Forza Italia ha fatto di tutto negli ultimi trentacinque anni per ridurre, ma che sono ancora alte. Vi leggo Vi leggo gli obblighi dei condomini a cui nessun proprietario si può sottrarre; attenzione, sono obblighi che condivido, perché molti di questi portano a una maggiore sicurezza, però è per far capire la situazione di vessazione della proprietà. Oltre alle tasse abbiamo la verifica sulla potabilità dell'acqua, l'obbligo di installare le valvole termostatiche, l'obbligo di installare contabilizzatori di calore, la verifica dell'amianto, la verifica biennale della messa a terra, la verifica biennale degli ascensori, la verifica del cancello elettrico del passo carraio, il certificato di prevenzione incendi. Avremo a breve da ragionare sulla trasformazione e quindi sulla direttiva delle case *green*. C'è il modello 770 del condominio. Molti Comuni, non avendo i soldi per farlo, stanno trasferendo anche delle competenze strane, come quella di tenere pulito dalla neve il marciapiede, che fino a prova contraria è pubblico, prospiciente i condomini. Ricordo poi il fascicolo di sicurezza del condominio.

chi mette a reddito gli alloggi non produce più reddito, cioè gli alloggi non sono più in grado, quando li affitti, di garantire una minima rendita. Oggi il proprietario è fortunato se va in pari rispetto a a tutte le cose che deve fare. Questo ha prodotto un aumento, a volte anche sconsiderato in alcune città, del costo per gli inquilini, quindi il costo degli affitti è aumentato: il proprietario deve pagare di più e cerca di rivalersi sugli inquilini. Quindi, questa è la situazione generale in cui noi inseriamo questo decreto-legge salva casa. Immaginatevi uno di questi proprietari,

Anche i notai hanno gradualmente aumentato i controlli che una volta non si facevano, perché il notaio certificava di avere davanti il signor A che vendeva al signor B, e che il signor A era proprietario dell'immobile. Oggi i notai devono fare una serie inenarrabile di controlli, che a volte fanno emergere problemi che fanno diventare quell'immobile, magari venduto dieci volte, non vendibile per l'undicesima

che non hanno potuto accedere a quel beneficio proprio perché abitavano in un condominio che aveva delle minime difformità, ma che con le normative di questo periodo, cioè precedenti al decreto-legge salva casa, non si potevano comunque sanare.

tende e verande c'è un'altra cosa che nessuno ha detto. Io sono un esperto di diritto condominiale, per cui mi permetto di citare questa parte, che è sempre poco citata. In Italia

Tra l'altro, il fatto di poter chiudere con vetrate parti attualmente aperte, di poter installare le tende cosiddette invernali non solo dà la possibilità di utilizzare degli spazi in più, ma va a creare un'ulteriore coibentazione rispetto alla fuga di calore, visto che un obiettivo che tutti ci poniamo è quello di diminuire il consumo energetico nei condomini.

e quindi va sempre a piazzarsi nella parte alta dell'appartamento. Abbassare il soffitto, sempre che (premesso ormai c'è scritto anche nel decreto-legge) siano rispettate tutte le norme igienico-sanitarie (quindi deve essere areato e abbastanza grande), fa risparmiare

bloccati, inondati: si parla di 4 milioni di pratiche. Ci sono ancora altrettante pratiche di condoni edilizi del passato ferme. Ci sono milioni di italiani che vogliono fare tutte le cose che vi ho letto e non le possono fare, sono in difficoltà. Nessuno ha parlato del fallimento dei condomini, ma ne parlo io. Il condominio non può fallire tecnicamente, ma nel momento in cui

Questi nuovi immobili, magari un po' più piccoli, permetteranno di andare in controtendenza rispetto all'aumento dei costi per gli inquilini, perché potranno essere messi sul mercato a un costo inferiore. Aiuteremo, così, le persone a non dover necessariamente presentare richiesta per una casa popolare, che non c'è in questo momento,

saluto il sottosegretario Morelli in rappresentanza del Ministero dei trasporti, ma dispiace non avere qui con noi il Ministro che tanto ha detto su questo provvedimento. provvedimento. Fedele alla prassi di questo primo anno e mezzo di Governo Meloni, il Senato oggi è riunito per votare quello che è stato ed è, a tutti gli effetti, un decreto elettorale. Lo è perché è stato annunciato poco prima delle elezioni europee, lo è perché, come tutto ciò che promettete in campagna elettorale, non risolve alcun problema. È servito solo a fare da megafono al vostro desiderio di apparire come impegnati a fare qualcosa di utile per il Paese, esattamente come avete fatto con l'altro decreto, quello che per finalità definirei gemello a quello che stiamo esaminando oggi. Mi riferisco al decreto liste d'attesa, annunciato come salvifica sferzata per il nostro sistema sanitario e dimostratosi esclusivamente fuffa sin da subito. Questo non perché ve l'abbiamo detto noi, ma perché ve l'hanno detto i vostri governatori. *(Applausi)*. Per raccogliere qualche consenso, quindi, chiamate un decreto salva casa, perché chiamarlo per quello che realmente è, cioè l'ennesimo condono, effettivamente non era cosa carina da fare. Ma la cosa più chiara è una, ovvero l'obiettivo, che non è risolvere le storture esistenti; l'obiettivo politico, quello vero, è il consenso in vista di una competizione elettorale. Il risultato, cioè questo provvedimento, è l'ennesimo pastrocchio di una maggioranza che non pensa certo a governare, perché ogni vostro provvedimento, ogni vostro decreto, ogni vostra iniziativa rappresenta la scusa per dare la colpa a quelli che vi hanno preceduto, come è successo poco fa, del resto. Ma veniamo al provvedimento nel merito. All'inizio la cosa ci faceva ben sperare, anche noi del MoVimento 5 Stelle ci siamo messi a disposizione per dare il nostro contributo, come dimostrano le proposte emendative depositate in particolar modo alla Camera, perché qui in Senato non è che ci abbiate dato dei grandi tempi per poter fare qualcosa, ma questa ormai è una prassi e lo sappiamo; è vostra abitudine e ci stiamo abituando. L'obiettivo da voi dichiarato con questo provvedimento doveva essere quello di migliorare la qualità dell'abitare nel nostro Paese, ma tra il dire e il fare, come al solito, c'è di mezzo il mare. Potete anche insistere, come state facendo, nel dire che non si tratta di un condono, ma la puzza del condono si sente lontano un miglio e si aggiunge al passaggio dal silenzio diniego al silenzio assenso, con la maggior maggior parte dei Comuni privi o carenti di risorse umane necessarie ad evadere migliaia di pratiche in soli quarantacinque giorni. Questo supera di gran lunga l'idea di una sanatoria della finestrella, come diceva il Ministro, e del piccolo abuso edilizio. Arrivate a sanare un po' di tutto, altro che piccole irregolarità. Leggete meglio il provvedimento di cui stiamo discutendo. Un conto sarebbe stato esaminare un provvedimento *ad hoc* che rivedesse davvero il testo unico dell'edilizia e tutte le norme sulla rigenerazione urbana. Ma chi vogliamo prendere in giro se nella Commissione 8a da mesi sono fermi tutti i disegni di legge depositati sulla rigenerazione urbana? È la volontà politica quella che vi manca che invece avete quando si tratta di andare a sanare condizioni che riguardano chi la casa già ce l'ha

e non certo alle variazioni essenziali che l'articolo 32 della legge n. 380 del 2001, il testo unico dell'edilizia, elenca chiaramente. Faccio l'elenco visto che comunque pare che questo punto non sia chiaro nemmeno a voi della maggioranza. Lettera *a)*, mutamento della destinazione d'uso; lettera *b)*, aumento consistente della cubatura della superficie del solaio; lettera *c)*, modifiche sostanziali di parametri urbanistico edilizi; lettera *d)*, mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito; soprattutto la lettera *e)*, violazioni alle norme vigenti in materia di edilizia antisismica. Dispiace aver sentito il commissario Castelli intervenire andando da tutt'altra parte e giustificare l'ingiustificabile di questo abominio che state mettendo in atto. È inutile che tergiversate e fate finta di niente. Con la vostra sanatoria - sì, chiamiamola così si regolarizzano anche fabbricati aventi forme e dimensioni diverse da quelli autorizzati, anche se non rispettano la normativa antisismica. In un Paese come l'Italia, caratterizzato da un territorio ad alto rischio sismico, che ancora conta il numero delle vittime prodotte da questi vittime prodotte da questi catastrofici eventi, voi favorite le costruzioni che non rispettano la normativa antisismica? È assurdo e davvero a stento trovo le parole per esprimere tutta la nostra contrarietà. Posso solo portare un esempio. Un edificio costruito negli anni Novanta, che rispetta le normative di allora, ma non rispetta quelle di oggi, può essere sanato senza colpo ferire. Magari fosse tutto qui e no, c'è dell'altro. Alla sanatoria sono interessati gli immobili sottoposti a vincolo storico, artistico e archeologico.

del paesaggio. Alla fine questo provvedimento è un altro regalo ben infiocchettato a quanti contano su di voi per riparare abusi e sotterfugi. Sempre nel merito del provvedimento appare evidente che il testo che avete proposto non risponde alle esigenze abitative; non riduce il consumo del suolo, non recupera il patrimonio edilizio, non riduce il carico delle delle amministrazioni comunali e potrei continuare. Queste erano le vostre premesse al decreto-legge. Queste misure semplificano la vita dei cittadini? No, la semplificano solo ad alcuni cittadini e a qualche scaltro immobiliarista. Questo provvedimento è un altro dei vostri capolavori. Colleghi della maggioranza e membro del Governo, nel nostro Paese ci sono 600.000 famiglie che hanno fatto domanda per una casa popolare. Quasi 200.000 rischiano il pignoramento della propria casa perché non riescono a pagare il mutuo; per non parlare poi degli sfratti che vedono 200.000 richieste, quasi 150 sfratti al giorno. Era questa l'emergenza da affrontare, a queste persone dovevate dare una casa, delle risposte e delle certezze. *(Applausi)*. Nel momento in cui noi discutiamo di questa roba è accaduto quello che è accaduto a Napoli, alla Vela Azzurra di Scampia.

che conoscete meglio. Ma noi, come MoVimento 5 Stelle, non possiamo lasciarvi fare, non possiamo lasciare che le nostre città affoghino nel cemento, senza il rispetto di *standard* urbanistici adeguati e di una eccellente qualità della vita degli italiani. Noi non possiamo abbandonare i funzionari comunali i funzionari delle Soprintendenze alle loro responsabilità, sovraccaricandoli di procedure e dando loro poco tempo per rispondere, invocando il silenzio assenso in nome della celerità, che finisce invece per violentare sempre più il nostro territorio, il nostro paesaggio e la nostra italianità. Concludo, Presidente, con una punta di amarezza per l'occasione che con questo provvedimento si è deciso di buttare alle ortiche. Capisco che dal vostro punto di vista appare logico, una volta definite le tasse il pizzo di Stato, continuare a dare una mano a chi è abituato a fare il furbo. Questo provvedimento è come gli altri, un altro mattone (per restare in tema)

Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, quando il Ministro aveva annunciato, durante un *question time*, che si stava preoccupando di fare questo decreto-legge per sanare qualche abuso, principalmente perché i notai non riuscivano a stipulare gli atti, e nello specifico ebbe a dire "non è possibile che ci sono case con tramezzature diverse rispetto ai progetti approvati, per cui bisogna ricorrere a una forma di recupero e di regolarizzazione", non vi nascondo che mi ero preoccupato, perché, se il nostro compito doveva essere così riduttivo, forse mi sentivo un attimino sminuito.

In quel momento, visto che i colleghi spesso ricorrono ai "Promessi sposi", ho immaginato il bravo che s'avvicinava a don Abbondio e gli sussurrava all'orecchio "questo matrimonio non s'ha da fare, né domani, mi sarei aspettato invece, dall'altra parte, un po' di interventi più costruttivi, un po' di interventi di contenuti. Oggi abbiamo cambiato un po' il *trend* in quest'Aula. Spesso ci accusate che la maggioranza non interviene; invece oggi, su dieci interventi, sette li fa la maggioranza e tre li fa l'opposizione. Ci saremmo aspettati invece più interventi, per cercare di capire in realtà cosa ci proponevate. Sento parlare di governo del territorio piuttosto che di edilizia. Generalmente sono abituato ad ascoltare e spesso riscontro o delle incoerenze fra di loro oppure delle inesattezze; ma io penso che sia le une che le altre scaturiscano da interventi fatti per partito preso. Chi mi ha preceduto, nella persona del collega Sigismondi, vi ha dimostrato che in 19 Regioni determinati provvedimenti che fanno parte di questo decreto-legge sono già in vigore e, di queste 19 Regioni, 12 sono di centrosinistra. Allora mi chiedo: perché nelle Regioni il centrosinistra prevede di fare questo tipo di attività in edilizia e, all'interno del Senato, lo stesso centrosinistra dice invece che queste cose non si possono fare? Mi nasce naturalmente qualche dubbio. Voglio rispondere a qualche collega, quando parla di governo del territorio. Lo sappiamo che oggi, nel 2024, quando parliamo di governo del territorio facciamo riferimento alla legge n. 1150 del 1942? Non c'è stato un aggiornamento di quella legge. È di questo che ci dovremmo preoccupare. Io sono componente anche della Commissione semplificazione e faccio parte dell'Intergruppo parlamentare Progetto Italia; con i colleghi ci stiamo occupando e preoccupando di rivedere questo testo del 1942. del 1942. Così come non è opportuno, nel 2024, parlare di edilizia facendo riferimento al DPR n. 380 del 2001: ventitré anni fa. In vent'anni penso che le città si evolvano. Quando, nel 1942, è stato fatto un piano, è stata fatta anche una legge. Quella legge, naturalmente, prevedeva l'infrastrutturazione, l'espansione dei territori, perché non esistevano le città. Oggi le città ci sono e, probabilmente, sono anche sovraffollate. Forse dovremmo prendere atto di questo. Forse dovremmo iniziare a pensare a una ristrutturazione, a una riqualificazione. Dovremmo pensare a qualificare i centri storici, quei centri storici che purtroppo si stanno abbandonando, prevedendo delle demolizioni con conseguente ricostruzioni, se veramente vogliamo dedicarci alla politica della casa e alla politica e alla politica del territorio. Io non capisco perché ci si accusi addirittura di non aver letto il testo. Io faccio una differenza tra cosa è leggere il testo e cosa, invece, è capirlo. *(Applausi)*. Dagli interventi che abbiamo ascoltato Dagli interventi che abbiamo ascoltato in Aula, mi rendo conto che, purtroppo, c'è qualcuno che non ha letto tanto per, perché se oggi mi si viene a parlare di condoni e di sanatorie, significa che non si capisce che cosa stiamo facendo. Mi farebbe piacere porre una domanda: cosa si sarebbe potuto fare ieri, piuttosto che oggi che stiamo discutendo il decreto? Ma secondo voi, un'opera difforme dal permesso di costruire non si sarebbe potuta sanare o condonare? Non è così, Non è così, perché un articolo del DPR sull'edilizia prevede che le opere non demolibili possono essere sanate. Per opere non demolibili, si fa riferimento a quelle opere che durante la demolizione possono creare nocumento alla parte sottostante. Però, come si possono sanare? Con una sanzione pecuniaria, pagando. Quindi, se paghiamo, possiamo sanare; se invece non paghiamo e diamo la possibilità di sanare senza pagare, non lo possiamo fare. se c'è contrasto con la normativa sui beni ambientali successivamente alla realizzazione dopo il 2004, quando subentra il decreto legislativo sui beni ambientali, non è possibile sanare. Però, se ricorriamo al danno ambientale, lo possiamo fare. E qui mi vengono in mente Totò e Peppino, quando facevano i falsari, che per loro era una questione di "lirica". Allora, se interveniamo sulle tasche dei contribuenti,

Penso che sarà difficile trovarla. Convengo, dunque, con il collega quando dice che dovremmo preoccuparci oggi per evitare domani di continuare a parlare di sanatoria. Dovremmo iniziare a studiare oggi qualche misura che ci dia la possibilità di controllare durante l'esecuzione dei lavori. Perché non attiviamo il controllo edilizio in forma stabile? Perché non prevediamo una sorta di stati di avanzamento durante le costruzioni, in modo tale che il controllo edilizio vada a verificare? Tanto basta verificare solo finché si crea l'involucro strutturale, perché dopo altri abusi non se ne possono fare. Di questo dovremmo iniziare a parlare. Questo decreto serve principalmente per cercare di chiarire e di fare un po' di chiarezza contro quella burocrazia che purtroppo non applica la norma, bensì la interpreta. Con troppa facilità negli uffici ci si sente dire addirittura che il parapetto di una copertura piana di altezza di un metro, necessaria per una questione di sicurezza, viene calcolata nell'altezza del fabbricato. Vogliamo parlare di risparmio del suolo? Allora consentiamo un'altezza libera nella realizzazione dei fabbricati, sempre mantenendo quei parametri urbanistici che determinano il volume da poter realizzare su quel lotto. Ma diamo un'altezza libera, in modo tale che si restringe la sagoma del fabbricato, si va in altezza e si recupera automaticamente del suolo. Come è pensabile che un pergolato ombreggiante realizzato su un tetto piano venga considerato tra le altezze? Ma quale altezza va a fare un pergolato ombreggiante? È di tutte queste cose ci piacerebbe parlare su di esse confrontarci. Io non sono solito dire: perché non lo avete fatto voi, visto che avete governato? Purtroppo, però, voi ci tirate per la giacchetta. L'unica cosa che siete stati capaci di fare è il RET, il regolamento edilizio unico i parametri, dove avete stabilito addirittura le definizioni dei parametri edilizi ed urbanistici. E lì c'è stato lo sfacelo: che significa che uno sporto di un balcone superiore a un metro e cinquanta viene calcolato nella superficie del fabbricato? Se il balcone è un metro e cinquanta piuttosto che un metro e sessanta, che cosa cambia? Che significa che se una veranda supera una metratura, in riferimento alla superficie utile dell'appartamento, viene considerata nel volume del fabbricato?

che oggi l'edilizia sia uno dei settori trainanti dell'economia locale, dell'economia italiana. Addirittura incide per una percentuale non indifferente sul PIL,

Tra noi e voi c'è una differenza sostanziale: noi ci preoccupiamo di tutelare chi legittimamente ha una casa, al contrario voi vi preoccupate e incentivate l'occupazione abusiva delle case.

mi sono fatto un'idea molto precisa dopo la discussione. Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato a capire che stiamo discutendo di un decreto-legge, però si vuole fare altro. Questo è il dato fondamentale. Si giustifica sostanzialmente l'intervento per la correzione di alcune particolarità, ma allo stesso tempo - mi pare che il senatore Rosso l'abbia posto in modo chiaro - il problema è il mercato mercato della casa. Ora, io non penso all'esproprio proletario anche perché sono padrone anch'io della mia casa, quindi faccio parte di quell'80 per cento di italiani che ha casa propria e se l'è sudata senza occupare niente, con i sacrifici suoi e della sua famiglia, suoi e della sua famiglia, quindi vorrei intervenire su questo elemento. Qual è la prima obiezione? Qual è l'urgenza di fare un decreto e addirittura di porre la fiducia? Avete la maggioranza.

si chiama B&B. Sapete tutti che nelle città non si trova più una casa in affitto. Lo sapete tutti. Non lo devo spiegare io.

per dare un immediato sostegno al fabbisogno abitativo che c'è, al recupero del patrimonio edilizio, un problema esistente, a ridurre il consumo di suolo, a intervenire sul contenimento energetico, a intervenire sulla questione della messa in sicurezza antisismica. Tutto questo non c'è. In questo decreto-legge non si parla di queste cose.

costruire, altro che non aumentare i volumi. Qui si aumentano enormemente i volumi. Basti pensare che da un *garage* un locale, questo è il dato fondamentale. Se però una casa è stata costruita prevedendo un *garage*, perché deve diventare un locale? Perché c'è un'esigenza? Certo che le esigenze ci sono, però attenzione, perché qui siamo di fronte a un condono

Ad esempio, ci sono 90.000 alloggi da risistemare. Provate per esempio a ragionare sulle

Se però vanno a studiare fuori e devono spendere 700-800 euro per una camera, non tutti possono permetterselo. Due operai o due impiegati che hanno un figlio o una figlia che va all'università, se una camera ha questo costo,

queste le cose che chiedono i cittadini e le cittadine, se vogliamo affrontare il problema. Se vogliamo dire che oggi c'è un mercato che chiede di avere queste cose, piccoli locali e roba di questo genere mordi e fuggi, benissimo. Se è questo, però, signori miei,

Tutto questo non interviene, come ho detto prima, sul contenimento energetico, perché non mi dite che se si trasformano un *garage* o un altro

di cui stiamo aspettando la rigenerazione, com'è stata definita, grazie anche ai fondi del PNRR, che spero potranno essere presto spesi grazie a una collaborazione, che sta avvenendo in maniera molto positiva, tra il Governo e le amministrazioni locali. Continuiamo a parlare di casa, che è un bene pur pur sempre associato a un concetto di potenzialità di investimento a livello economico e finanziario; è un bene il cui valore si mantiene sempre abbastanza stabile nasce la definizione di bene rifugio. Ancor più la casa è però il luogo dello sviluppo personale, relazionale e anche affettivo; è un luogo strettamente personale, perché è essenziale per uno dei bisogni principali dell'essere umano. C'è quindi da rimanere indignati al ricordo di quei Governi tecnici che, guarda caso sempre sorretti dalla sinistra, dagli anni Novanta hanno deciso di incidere su questo bene, considerandolo il salvadanaio non delocalizzabile da aggredire con priorità su ogni altra azione politico-economica. Ben diverso è il fronte che oggi invece, per coerenza, grazie alla Lega e al ministro Matteo Salvini, stiamo concretizzando con un *corpus* di norme che definirei di agevolazione semplificatoria, un'azione di valorizzazione patrimoniale, com'è stato detto da molti esponenti del centrodestra che sono intervenuti nel corso di questa discussione generale. Di ciò hanno avuto immediata contezza proprio le categorie professionali (che ho sentito poco ricordare da parte delle opposizioni), che invece oggi plaudono al via libera al decreto-legge salva casa, fortemente voluto dal vice *premier* Matteo Salvini. Tra questi possiamo citare moltissimi interventi, ma ne ho scelti alcuni che sicuramente interesseranno anche gli amici dell'opposizione. Tra i tanti sostenitori di questo testo c'è Irene Sassetti,

carica che rende le dichiarazioni rilasciate ancor più interessanti. La consigliera dice che si tratta di un intervento per razionalizzare le norme e superare le difformità minori che non intaccano minimamente la sicurezza dell'edificio, quindi è un testo che non va demonizzato. Sono parole che destano una buona meraviglia, ma voglio raccogliere anche un'altra testimonianza, sempre dal mio territorio, significativa di un contesto immobiliare particolarmente gravato dalle irregolarità costruttive. Il geometra Dario Cerrai, presidente del Collegio dei geometri di Livorno, ha affermato alla stampa che si tratta di una misura necessaria, poiché serviva un provvedimento che aiutasse la circolazione dei beni. Con la doppia conformità il mercato immobiliare si è infatti bloccato e lo hanno confermato diversi tra i colleghi che sono intervenuti. È stato stimato che, prima delle modifiche apportate alla Camera al testo voluto dal vice *premier* Matteo Salvini, solo nella città di Livorno si stimavano 4.000 potenziali domande che avrebbero potuto essere avviate già solo con le norme originarie di questo testo. testo. Lo scopo del decreto, come confermato dagli operatori del settore, è quindi quello di intervenire sulle violazioni di minor peso per non pregiudicare la commerciabilità degli immobili e va detto che il nostro patrimonio edilizio ne aveva davvero bisogno. Sono molte le difformità per le quali il piccolo proprietario pensava di essere in regola, ma rispetto alle quali, a seguito di relazioni di conformità, si è accorto di non esserlo, a causa magari di finestre o di pareti. di pareti. Sembra assurdo dirlo, ma l'immobile in quel momento diveniva invendibile, perché la norma non consentiva di procedere con il criterio della doppia conformità. È sembrata una piccola rivoluzione copernicana, ma devo dire che avercela fatta è stata una cosa straordinaria e da ora in poi questo sarà un problema risolvibile grazie allo stato legittimo stabilito dal titolo abilitativo che ne aveva previsto magari la costruzione oppure quello che ne ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio. devo dire che il mio Gruppo è assolutamente contento del fatto che resti un impianto, a seguito del lavoro svolto dalla Camera dei deputati, frutto di un confronto e foriero di ben sette modalità di sanatoria e regolarizzazione, su difformità parziali, variazioni essenziali, tolleranze costruttive ed esecutive, legate ad aspetti igienico-sanitari, varianti *ante-*1977 e difformità non contestate in fase di rilascio dell'abitabilità; inoltre, deroghe ai criteri fissati dal Ministero della sanità nel 1975, dichiarando agibili immobili con altezze di 2,4 metri e di superfici di 20 metri quadri per monolocali e 28 per bilocali. Mi ha

vorranno avviare grazie alle norme volute dal ministro Salvini. Un altro appunto circa le accuse di voler andare a realizzare un condono edilizio: il desiderio, ad esempio, di esercitare in maniera esclusiva poteri che l'articolo 117 riconosce in maniera concorrente a Stato e Regioni viene proprio dalle Regioni di sinistra. La mia Regione, la Toscana, è stata quella che ha avuto i più esemplari contenziosi in sede di Corte costituzionale proprio in materia di condono *extra ordinem*. Voglio ricordare, tra tutte, la famosa sentenza n. 233 del 2015, nella quale la materia del contendere era costituita da una normativa regionale voluta dalla Regione Toscana amministrata dal PD, nella quale si andavano addirittura ad elidere e ad attenuare gli obblighi di vigilanza comunale per la repressione degli abusi che la Corte costituzionale ha ritenuto correttamente essere una materia di competenza esclusivamente statale in forza del testo unico degli enti locali. Vorrei ricordare però anche i tentativi di intervenire, sempre da parte della Regione Toscana, sulle sanzioni per opere ed interventi abusivi edilizi anteriori alla

Per gli amici della Regione Toscana, ben venga che presto anche questa competenza in maniera di territorio potrà essere esclusivamente richiesta in esercizio da parte delle Regioni; probabilmente, gli amici di sinistra risolveranno i loro grattacapi relativamente alla volontà di sanare qualcosa. In conclusione, vorrei ricordare alla nostra maggioranza che questo è un grande lavoro, nato appunto dalla condivisione di principi liberali e libertari, che riguardano un bene prezioso che gli italiani hanno costruito. L'amico e collega espressione della sinistra ha voluto coraggiosamente ricordare come gli italiani abbiano fatto sacrifici per acquistare una casa, non l'abbiano voluta occupare, ne siano orgogliosamente proprietari ed abbiano assolutamente il diritto di esercitare tutte le loro signorie, permesse dai codici e dalle leggi dello Stato su quell'immobile. In questo condivido il pensiero del collega Magni, che viene da sinistra, ma è espressione di una corretta, intellettuale e pulita concezione della proprietà privata, diversamente da alcuni suoi colleghi, che invece ne hanno un'idea ben diversa. *(Applausi)*.

Il collega Rosa, a cui riconosco onestà intellettuale, ha detto all'inizio di questa discussione che nel breve tempo che abbiamo avuto abbiamo fatto una discussione generale e discusso emendamenti. Ieri in Commissione è stata depositata la legge e dopo due ore dovevano essere depositate le proposte emendative: abbiamo atteso che la Commissione fosse riconvocata più volte per discutere il fascicolo degli emendamenti, ma non si è discusso di mezzo emendamento. Per essere onesti fino in fondo, noi non abbiamo discusso di questa legge. È questo il punto. Ormai c'è un monocameralismo a cui in particolare noi come Senato ci siamo adeguati: la discussione si è svolta alla Camera, è stato solo un esercizio formale, abbiamo solo depositato carta con inchiostro e consegnato all'Aula adesso una discussione che in realtà si è già fatta altrove. Avevamo invece proprio bisogno di fare una riflessione che componesse tutto il processo legislativo intorno al tema della casa. Rigenerazione urbana, ricostruzione (intesa anche come codice della ricostruzione), contrasto al consumo del suolo, *bonus* edilizi, affitti brevi, edilizia popolare: sono solo alcuni dei tanti temi che viaggiano su testi e leggi diversi, che non parlano tra di loro e la provvidenza dovrebbe comporre, ma che invece il Parlamento, la politica e il potere esecutivo con quello legislativo dovrebbero comporre in un'unica visione di diritto all'abitare, in un'unica riflessione. Come ha detto il senatore Rosso, questo provvedimento ha incontrato il favore dei corpi intermedi e dei rappresentanti di interessi. A noi non risulta, forse parliamo con soggetti diversi: dall'ANCE ai sindacati, compresa tutta la filiera della costruzione,

con questa filiera e registrato un profondo disagio. Rimettiamo le cose in ordine. Intanto, è consuetudine nel confronto parlamentare di questa legislatura un eccesso del ricorso alla decretazione d'urgenza come mezzo di cui il Governo abusa per emanare provvedimenti normativi in ogni materia. Siamo ormai al sessantottesimo decreto-legge. Anche questo, come quasi tutti gli altri, è privo dei fondamentali presupposti di necessità e urgenza previsti dalla Costituzione, lo abbiamo detto. È ormai chiaro che all'interno del Governo c'è la volontà di snaturare nel profondo il dibattito parlamentare e piegarlo a tempi e modi congeniali ai propri interessi di parte. Il tema in questione, la casa, non è solo una grande emergenza per un'ampia parte della popolazione, ma anche il più grande patrimonio per le famiglie e un *asset* strategico per l'economia del Paese, se reso oggetto di avvedute politiche pubbliche. Come in altri campi, però, è proprio questo che manca, una strategia e un piano di rilancio del bene casa, di cui il decreto-legge in conversione rappresenta come non mai un esempio negativo, carente, senza visione e frutto di una cultura politica che chiama salva casa un provvedimento normativo che è una caotica e ampia deregolamentazione. Quest'affermazione non è il frutto di un approccio ideologico a quanto stiamo discutendo. Non ve ne sarebbe alcun motivo, né convenienza politica, Non può essere questo il terreno di scontro dialettico su cui far prevalere ragioni di ordine ideologico, motivo di pregiudizio politico, né ottuse chiusure nel merito. Penso ad esempio - e lo dico in via preliminare, per sgomberare il campo - che il miglior modo per tutelare regole e legalità sia certamente quello di semplificare i cavilli burocratici e che il miglior modo per far crescere una cultura del rispetto delle regole sia quello di andare incontro alle persone. Non penso dunque a un sistema che in materia urbanistica ed edilizia faccia della vigilanza e della sanzione le uniche modalità di esercizio delle prerogative affidate agli enti preposti. Tuttavia, il testo che siamo chiamati a discutere e il dibattito parlamentare, sia quello in occasione dell'approvazione alla Camera, sia quello che sta si sta svolgendo qui, restituiscono con chiarezza i motivi di fondo della norma e degli obiettivi più o meno reconditi che abbiamo di fronte. Diciamoci la verità: questo provvedimento si preoccupa soltanto di sostenere la rendita immobiliare e di permettere l'immissione sul mercato di immobili che finora non avevano la possibilità di starci. Lo fa introducendo modifiche al DPR n. 380 del 2001, per liberalizzare le categorie di interventi nella cosiddetta edilizia libera, semplificare la documentazione attestante lo stato legittimo degli immobili, allargando le maglie della disciplina dei cambi di destinazione d'uso non solo per singole unità immobiliari, ma addirittura per interi immobili, ampliando la disciplina di acquisti o alienazioni per opere acquisite dal Comune ed eseguite in assenza di permesso di costruire e poi avventurandosi nella delicata materia delle tolleranze costruttive e del superamento della cosiddetta doppia conformità per le aree sottoposte a vincolo storico, ambientale e persino di pericolo idraulico e idrogeologico. Pur volendo forzosamente riscontrare che in taluni sporadici casi tra quelli citati possano esserci elementi di semplificazione utili a risolvere problematiche stratificate nel tempo e che rendono la vita difficile a famiglie destinatarie di piccole eredità immobiliari e a piccoli proprietari che magari intendono alienare modeste proprietà e non possono farlo per cavilli formali, resta inequivocabile l'impianto di fondo che avete voluto per questa norma: una generale e indiscriminata sanatoria, che consentirà grandi affari e grandi guadagni ai detentori di ingenti patrimoni. D'altronde, se consentite di rendere abitabili alloggi con un solo vano di 20 metri quadri - come diceva il senatore Irto - con altezza di due metri e quaranta, sanando sottotetti e cantine; se aumentate le percentuali delle tolleranze costruttive e le difformità per altezze, distacchi, cubature e superfici delle case fino a 60 metri quadri; se consentite lo scostamento per difformità rispetto al progetto approvato per cento; se consentite di cambiare destinazione d'uso degli immobili, infine, state effettivamente aprendo a un generalizzato provvedimento di sanatoria. Tale provvedimento incentiverà il fenomeno d'impoverimento residenziale delle aree urbane e dei centri storici, moltiplicando il fenomeno degli affitti brevi e turistici. Su questo fronte il provvedimento alla Camera (perché qui è stato inutile), introducendo misure di rafforzamento dei poteri comunali attraverso regolamenti e strumenti urbanistici, ma ogni nostra proposta è stata respinta, alla faccia della sussidiarietà istituzionale e del vostro altalenante spirito autonomista. Al cospetto di tutto questo, dove sono invece gli attesi e sacrosanti provvedimenti, questi sì improcrastinabili, per il sostegno agli affitti, per rifinanziare il fondo affitti e morosità incolpevole, ovvero i provvedimenti urgenti per affrontare la carenza di case per studenti e studentesse e di alloggi di edilizia residenziale pubblica per le famiglie a basso reddito? Non può essere condivisa né tollerata l'argomentazione per la quale questo provvedimento sarebbe utile all'emersione dell'abusivismo e di tanti immobili fantasma. Anche qui - diciamoci la verità - abbiamo avuto nel recente passato una misura che ha consentito un'ampia azione di emersione. Proprio la vituperata scelta del superbonus al 110 per cento bisogna dire con onestà, soprattutto tra le file della maggioranza - ha portato alla luce migliaia di immobili: la più grande opera di recupero di evasione ed elusione fiscale sul patrimonio immobiliare, garantita e sostenuta da politiche pubbliche di incentivo alla messa in sicurezza e all'adeguamento energetico. Sono decine di migliaia gli accatastamenti di immobili che erano nascosti al fisco, decine di migliaia le SCIA in sanatoria depositate negli uffici tecnici dei Comuni e decine di migliaia i depositi negli uffici del Genio civile che hanno riportato alla luce un patrimonio immobiliare sconosciuto allo Stato, e sono milioni di euro quelli recuperati all'erario e alle casse dei Comuni per mezzo della tassazione di immobili fino a pochi anni fa inesistenti. Sarebbe stata questa la giusta strada da seguire, se si fosse voluto costruire un vero provvedimento salva casa. Modificare, certo, magari nel profondo la normativa dei *bonus* edilizi e magari costruire un nuovo provvedimento organico che restituisse coerenza alle stratificazioni normative accumulate negli anni, capace di coniugare adeguamento energetico, sostegno alle imprese, lavoro di qualità e anche emersione e regolarizzazione degli abusi, per per mezzo di semplificazione normativa. La strada imboccata è invece un'altra ed è chiarissima: *deregulation*, incentivo alla rendita, un liberi tutti che favorisce le speculazioni e non si occupa dei veri problemi, tutto questo in un clima di profonda divisione all'interno della maggioranza: bisogna dire anche questo. Abbiamo assistito a un travagliato dibattito alla Camera, che ha partorito addirittura emendamenti solo nelle fila della maggioranza e ha lasciato sul campo la vicenda Milano-Cortina come vittima immolata alle incomprensioni interne di un Governo diviso. È andato in onda un pessimo spettacolo, che non ha aiutato a migliorare, emendare e correggere un provvedimento profondamente sbagliato e dannoso, da parte di una maggioranza e un Governo ormai sempre più divisi e che, su questo provvedimento, hanno dato ampia dimostrazione delle lacerazioni crescenti. Purtroppo, a farne le spese, anche in questo caso, è e sarà il Paese.

69 del 2024, che appunto interessa il tema della semplificazione edilizia e urbanistica, è un provvedimento per noi molto importante, che si inserisce in un'idea complessiva, perseguita da questa maggioranza e da questo Governo, di dare più attenzione alle politiche del territorio, sicuramente trascurate e tralasciate negli ultimi anni dal Parlamento, che se n'è occupato solo in relazione a emergenze legate alle fragilità e alle problematiche del nostro territorio. Pertanto, iniziamo con questo provvedimento, perché riteniamo urgente partire dalla rimozione di quegli ostacoli burocratici che limitano la fruizione e il godimento di un bene essenziale e primario come la casa, che è una ricchezza non solo economica, ma morale e culturale dell'Italia che è stata di fatto danneggiata da una burocrazia che ci saremmo aspettati di individuare insieme, in occasione di questo provvedimento, come avversaria. Invece, da parte dell'opposizione, si è scelto di argomentare diversamente: legittimamente, ma in modo ampiamente confutabile. Infatti, le modifiche al testo unico dell'edilizia che ci accingiamo ad approvare,

il recupero dei sottotetti qualcuno l'ha definito una misura scandalosa. Invece, è una norma di buonsenso che, tra l'altro, fa salva la normativa regionale, che può ampiamente intervenire rispetto al tema idrogeologico e quindi valutare la compatibilità di questo tipo di interventi. Con gli interventi sull'edilizia libera, stiamo parlando di consentire ai cittadini la chiusura di vetrate e tende. Parliamo di questo e qualcuno ha il coraggio di gridare allo scandalo e alla sanatoria.

gli altri colleghi di Fratelli d'Italia in particolar modo, si riferiscono a edificazioni realizzate prima della normativa per la quale poi quegli interventi sono stati contestati.

per alcuni partiti di opposizione valga solo quando questi interventi che ci chiede l'Europa penalizzano i cittadini; quando invece riguardano un beneficio, una facilitazione o una semplificazione, diventano interventi scandalosi. il declassamento di alcune variazioni a non essenziali; l'incremento delle sanzioni, quando la demolizione degli immobili abusivi non è possibile; le tolleranze costruttive portate entro il 2 per cento (pensate che percentuale scandalosa, che determina un condono); la disciplina di interventi in parziale difformità e, soprattutto, come hanno sempre detto molti dei colleghi di maggioranza, il superamento della doppia conformità in caso di parziale difformità, che giustamente per i cittadini che non si sono trovati alle prese con questo tema può non significare nulla, ma per molte famiglie è stato un incubo, per la burocrazia e causa dell'impossibilità di disporre di un bene come la casa, come il diritto con dovrebbe consentire e consente.

da questo punto di vista è importante che sia stata sancita in modo chiaro dal commissario alla ricostruzione, il senatore Castelli, l'assoluta falsità di qualsiasi riferimento al fatto che non dovrebbe più essere valida la normativa antisismica dopo questo provvedimento, grande *fake news* che ovviamente è stata ampiamente rispedita al mittente.

che siamo di fronte a norme che aiutano e supportano le famiglie, spesso ostaggio della burocrazia, e immettono nel mercato immobiliare abitazioni che erano di fatto sequestrate dalla burocrazia stessa.

Sono inoltre norme che favoriscono l'utilizzo dell'esistente, perché qui parliamo spesso di rigenerazione urbana. Discuteremo e stiamo discutendo, proprio qui in Senato, di rigenerazione urbana, ma per per poter limitare il consumo di suolo bisogna ovviamente valorizzare e liberare il patrimonio esistente dai vincoli e dai lacciuoli burocratici, altrimenti sono soltanto *slogan*. Qui non c'è nessuna sanatoria, quindi: l'unica cosa che si sana sono irregolarità formali e non sostanziali che hanno, in alcuni casi, rovinato la vita di intere famiglie. si rimuovono incertezze giuridiche e si afferma con più chiarezza lo stato di legittimità. Questo provvedimento corrisponde quindi a una visione che vuole uscire dalla confusione tra il sacrosanto rispetto della legalità e la burocrazia. Ci fa anche un po' sorridere il richiamo alla legalità da

è si è allontanato o vicende del genere (questo tipo di interventi viene anche difeso politicamente). Insomma, credo che il richiamo alla legalità lasci il tempo che trova.

di qualche legittimo proprietario, sappia che in quella casa non continuerà a stare in modo abusivo. Questo provvedimento importante non sarà un *unicum* - a proposito dei grandi temi da affrontare in questa legislatura e nel futuro - sul tema dell'urbanistica. Abbiamo parlato di rigenerazione urbana, ci sono provvedimenti in merito in Senato. Io credo che si potrà fare un confronto serio, ampio e partecipato alta, è quella di codificare un nuovo modello di urbanistica che riconnetta l'uomo al suo ambiente naturale e che lo faccia in modo serio. Ovviamente, abbiamo espresso tutti costernazione, sgomento e dolore per quello che è accaduto a Scampia, ma da molti anni sosteniamo che di fronte ad alcune realtà urbanistiche ci sia ben poco da rigenerare e si debba portare avanti il criterio della sostituzione edilizia, della demolizione e della ricostruzione.

con l'edificazione di altri mostri di cemento figli del turboliberismo e del turbocapitalismo. Comunque sono entrambe facce della stessa medaglia che noi dobbiamo andare a rimuovere per dare vita a un nuovo rinascimento urbano, per mettere al centro una nuova idea una nuova idea dell'abitare. Alcuni dogmi, come quello della città dei quindici minuti, ci convincono anche poco, perché a volte possono diventare un paravento per far diventare quella città e i

Queste sono sfide sicuramente importanti. Dobbiamo tornare quindi a una identità precisa dell'abitare, ma si parte dalla base: si parte dalla casa, quel bene

mettere in atto e lavorare con tutte le forze che abbiamo affinché possa essere il nostro *habitat*, il luogo dove ci possiamo riconnettere alla nostra identità, alla nostra cultura, ai luoghi dove viviamo. Per questo ci dobbiamo impegnare.

autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 1197, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. nuova finestra"). La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati. Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo,

e, per le dinamiche parlamentari, un abuso dell'utilizzo della apposizione della questione di fiducia, che consente un risparmio in ordine di tempo nella trattazione dei provvedimenti. Nessuno di noi è scevro da responsabilità in questo: è successo - come dicevo - negli ultimi vent'anni con tutti i Governi. Certo è che questo Governo sta battendo qualsiasi *record*. Nel frattempo, però, è intervenuta anche una modifica regolamentare in questo ramo del Parlamento, che consente in modo evidente di affrontare un provvedimento anche con l'urgenza che è caratteristica intrinseca dei disegni di legge di conversione in legge dei decreti-legge, che sono ovviamente per loro natura urgenti in quanto soggetti a potenziale scadenza della loro efficacia. Negli stessi tempi con cui si converte un decreto-legge, con la fiducia si può ragionare in Commissione, presentare emendamenti, spesso anche con il contributo delle opposizioni. Nell'ultima Conferenza dei Capigruppo - come sa bene il ministro Ciriani - su questo provvedimento le opposizioni si erano impegnate a presentare un numero limitatissimo di emendamenti per poter fare una discussione più ampia in Aula; più ampia significa qualche ora in più, ma per entrare nel merito dei singoli punti del provvedimento. il fatto che ci sia l'esigenza di avere il parere della Commissione bilancio rispetto a un provvedimento che nasce per non essere modificato, bastava che la Commissione bilancio - come fa molto spesso esprimesse un parere contrario per mancanza di relazione tecnica su tutti gli emendamenti delle opposizioni. Non c'erano emendamenti potenzialmente assentibili e approvabili. Quindi il ricorso in quest'Aula alla questione di fiducia è legato esclusivamente a motivi politici, al timore che il Governo ha nei confronti della propria maggioranza (e

Nel solco del mio intervento precedente molto rapido e cercando di approfondire alcuni aspetti, questo provvedimento contiene alcuni elementi certamente degni di attenzione e che pongono alcuni rimedi a oggettive criticità che persistono nella compravendita degli immobili e nel presentare un progetto di ristrutturazione di un immobile. È chiaro che lo stato legittimo è elemento essenziale della presentazione di un nuovo progetto. Pertanto, guardando alcuni degli elementi del decreto-legge non mi spaventa particolarmente il tema delle tolleranze. Non è particolarmente critico, anche se fatto in un modo - a mio avviso - troppo ampio, il tema del cambiamento di destinazione d'uso. al recupero dei sottotetti, vivo in una Regione che nella legge regionale ha già previsto sostanzialmente quello che oggi dispone il decreto-legge, e, se applicato con buon senso, può dare una risposta ad alcune esigenze abitative; il tema dello stato legittimo viene affrontato in uno dei modi possibili, ma sicuramente è un tema che viene affrontato. Tuttavia, intravedo alcune criticità piuttosto profonde rispetto al tema della doppia conformità.

portare il Governo, anche con un disegno di legge di iniziativa governativa, a consentire alle Camere di realizzare un percorso più ampio di discussione.

ho ben contezza di quale sia la complessità delle norme in tema di edilizia e urbanistica. Proprio per questo, però, una reale semplificazione doveva partire da una riscrittura del testo unico, con qualche tempo in più. Ma, se c'è la volontà politica, le Aule hanno sempre dimostrato di poter affrontare i temi nei tempi che servono alla discussione, ma anche all'approvazione dei provvedimenti. Ma veniamo a quello che qualcuno nell'intervento precedente ha citato come *fake news.* La *fake news* è quella che ha dato il commissario, persona che stimo, ma che - mi dispiace - ha citato solo un pezzo della verità. È vero, in caso di variazioni essenziali o di variazioni al progetto assentito che abbiano a che fare con la struttura dell'edificio, il tecnico può e deve valutare la corrispondenza dell'intervento anche rispetto alle norme tecniche sulle costruzioni ad oggi. Ma questo è vero soltanto per le aree non a bassa sismicità. però non significa che sono aree non sismiche, perché dal 2003, con la revisione della classificazione sismica, tutto il territorio italiano è zona sismica a bassa, media, alta o altissima pericolosità. Cambia l'accelerazione di progetto che si utilizza nel calcolo della risposta sismica di un fabbricato, che va da 0,05g, nel caso di bassa sismicità, a 0,35g, in zona sismica 4, che è la più alta. Faccio un esempio. In un territorio a bassissima sismicità non è più possibile aprire un foro in una parete perimetrale portante - come si faceva fino al 2008 - mettendo un architrave progettato alle tensioni ammissibili e aprendo il foro: bisogna garantire una risposta sismica della parete identica prima e dopo l'apertura del foro e ciò obbliga a una cerchiatura del foro finestra. Questo non verrà più valutato nelle variazioni essenziali di quelle zone che sono a bassa sismicità, perché la norma non lo prevede. Questo è un rischio per il Paese in oltre il 50 per cento del territorio italiano che è a bassa sismicità. Quindi, in tutte quelle parti del Paese che sono più del 50 per cento delle aree d'Italia a bassa sismicità, chi ha aperto quattro fori finestra progettandoli con le norme tecniche *ante* 2008 e ha fatto una variazione essenziale al proprio progetto non vedrà nessun tecnico abilitato valutare la risposta sismica di quel fabbricato, anche se con una intensità sismica molto limitata, pari a 0,05 g. Quindi, dire che dal punto di vista della sicurezza sismica nulla cambia è una *fake news*. O non lo si è capito o si fa finta di non capirlo. E dal punto di vista politico mi sarei aspettato una maggioranza che brindava all'aver introdotto una fattispecie di condono, perché in fondo è questa la postura di questa maggioranza dal punto di vista sia fiscale che edilizio. Invece, quasi nascondete quello che state facendo e non ne capisco la ragione. In fondo questo tipo di semplificazioni era oggetto anche del programma elettorale del centrodestra. È quasi come se la maggioranza si vergognasse di quello che sta facendo su questo punto. punto. Non ho sentito dire nessuno - come dicevo prima - che con le modifiche introdotte alla Camera la realizzazione di un piano in più, che non mi sembra una variazione di poco conto, come una paretina spostata

È del tutto evidente che la corrispondenza urbanistica ad oggi porta a un vantaggio urbanistico. È chiaro che i piani regolatori sono sempre stati i piani di sviluppo dell'attività edilizia, hanno sempre portato in aumento gli indici di cubatura e di edificabilità delle varie zone omogenee, mentre c'è stata una forte restrizione sulla parte edilizia, sia per le norme impiantistiche, sia per quanto riguarda le norme sismiche. E, quindi, aver sganciato in questo modo la doppia conformità il vero pericolo, perché ci siamo occupati della parte sismica, ma c'è tutta la parte impiantistica che segue esattamente la stessa razionalità. La nostra preoccupazione è che vi sia una parte del patrimonio edilizio di questo Paese che viene, sì, sanata, ma con un pericolo per la collettività e questo francamente non credo si possa accettarlo. Un ultimo passaggio svolto sulla questione dei vincoli e in qualche modo su una maggior tutela dei beni sottoposti a vincolo culturale, ambientale e paesaggistico. Anche da questo punto di vista, posso condividere il fatto che questo è un Paese in cui troppo spesso la tutela in qualche modo si è spostata sull'impossibilità a fare. Ma non è con le deroghe che riusciamo a raggiungere l'obiettivo di tutelare il patrimonio, che è necessario tutelare senza vincolare eccessivamente quel patrimonio che non ha senso tutelare. Intanto, la nostra cultura di conservatoria ha consentito oggi al nostro Paese di avere il patrimonio di beni culturali più ampio in tutto il mondo: i beni culturali di questo Paese sono superiori alla somma di tutti gli altri del resto del mondo proprio per questo nostro approccio di conservazione. Ma, se vogliamo ragionare su come migliorare il rapporto tra la conservazione dei beni e la necessità di operare sul patrimonio edilizio, dobbiamo modificare in modo strutturale le norme e non prevedere in ogni decreto delle deroghe. Anche questo è un lavoro certo più difficile, più complesso e più lungo.

"Il link apre una nuova finestra") *(PD-IDP)*. Signora Presidente, onorevoli senatrici e senatori, siamo di nuovo qui a intervenire contro la scelta scellerata di questo Governo di mettere la fiducia sulla conversione del decreto-legge. Siamo ancora qui a ribadire che questo modo di fare riscrive la natura stessa del Parlamento da luogo del processo legislativo a un mero organo di ratifica. In questo caso c'è anche di peggio e non possiamo non sottolinearlo. Il decreto-legge in esame ha concluso l'*iter* alla Camera diventando tutt'altro rispetto a quanto votato in Consiglio dei Ministri: un processo di allargamento delle norme e delle sanatorie che richiedeva un confronto vero e approfondito proprio in quest'Aula. Insomma, signor Presidente, mi verrebbe da dire che siamo stanchi e stufi di dover ripetere sempre le stesse recriminazioni davanti al comportamento di un Governo che sente di poter scavalcare il Parlamento. È semplicemente una vergogna, perché si riducono le istituzioni a cassa di risonanza dell'Esecutivo e si usa lo strumento della fiducia per accelerare i tempi e fare leggi in modo frettoloso;

le polemiche e i conflitti interni alla maggioranza; conflitti che abbiamo visto anche alla Camera con la presentazione di oltre 300 emendamenti da parte delle forze di maggioranza. Nel caso del decreto casa l'azzeramento del confronto e del voto sugli emendamenti è particolarmente grave, perché non ci consente di poter presentare proposte alternative a un testo come uscito dalla Camera dei deputati, che si presenta come la *summa* della deregolamentazione in ambito urbanistico; via ogni paletto, ogni parere o vincolo. Benvenuti nell'era del silenzio assenso che supera perfino ogni vincolo paesaggistico. Signora Presidente, mi sono letta con attenzione il testo di legge. Da ex assessore all'urbanistica e al recupero del patrimonio edilizio della città di Pisa, penso di conoscere bene i tanti problemi ancora irrisolti in questo settore e mi aspettavo sinceramente che si potesse compiere qualche passo in avanti. Ecco, prima di entrare nel merito degli articoli di legge, svelerò il finale del mio intervento. Questo provvedimento non risolve nulla e aggrava la situazione: nulla sul recupero del patrimonio edilizio esistente; nulla sul contrasto all'abusivismo edilizio e meno di nulla sul sostegno finanziario ai Comuni per far rispettare le regole e procedere nelle demolizioni; nulla sulla rigenerazione urbana, i cui fondi contenuti nel PNRR sono stati già irresponsabilmente tagliati da questo Governo; nulla sul diritto alla casa che oggi è vietato da politiche irresponsabili, come il taglio dei contributi all'affitto e per la morosità incolpevole; nulla sulla questione dei *bed and breakfast* che stanno invadendo i centri storici delle grandi città italiane. Allora cosa contiene questo decreto-legge di così urgente da giustificare l'azzeramento del confronto parlamentare e l'ennesima fiducia? Veniamo alle norme contenute nel testo che ci fanno gridare allo scandalo perché ribaltano i principi di legalità e, in alcuni casi, anche di costituzionalità, come abbiamo detto questa mattina. Siamo in presenza di una vera e propria sanatoria mascherata. Non ci sono altre parole per dirlo. Pensate alle norme che abbassano a 20 metri quadri la soglia per i monolocali e che abbassano - son cumulative queste due possibilità le altezze minime a 2,40 metri. Cosa significa? Questi loculi saranno appartamenti a tutti gli effetti e tutti i garage d'Italia e anche i sottotetti diventeranno appartamenti. Fermiamoci un attimo su questo, perché stiamo dando il via libera alla possibilità di far vivere una persona in 20 metri quadrati. Pensiamo a quello che è successo durante il Covid, alla pandemia e a come abbiamo vissuto chiusi dentro l'abitazione; pensiamo anche che avevamo detto che dovevamo apprendere quella lezione. Oggi invece vi presentate con delle norme che peggiorano una situazione già da correggere.

L'aspetto più grave è sicuramente l'eliminazione della doppia conformità e del limite dei novanta giorni, trascorso il quale scatta il meccanismo del silenzio assenso sulle domande di accertamento di conformità degli interventi edilizi. Eccola la vera e propria sanatoria. Proponete modifiche come se non fossero chiari i numeri dell'abusivismo edilizio in Italia. Durante le audizioni alla Camera Legambiente ha portato dati chiarissimi: solo nel 2022 il numero degli abusi edilizi è salito del 9,1 per cento, un fenomeno tutt'altro che in via di eliminazione. Il 42 per cento delle abitazioni è al Sud ed è stato costruito con abusi. È una situazione drammatica, insostenibile. E voi venite in quest'Aula, con queste nuove leggi, e ci chiedete anche di azzittirci, mettendo la fiducia. È semplicemente immorale. Avete addirittura introdotto il principio del silenzio assenso nelle aree vincolate, quelle dove ancora oggi insiste il principio dell'autorizzazione paesaggistica. Qui non siamo nel campo dell'etica, di norme sbagliate e inaccettabili: qui si apre un conflitto anche costituzionale. Introducete queste norme cancellando anche l'obbligo di ispezione dell'Ufficio di igiene e sicurezza; d'ora in avanti basterà una perizia asseverata di un tecnico. Dico questo perché molte delle semplificazioni contenute nel testo avranno come conseguenza l'aumento sconsiderato del lavoro presso gli uffici Ma se io istituisco il principio del silenzio assenso e poi concentro i controlli in capo al Comune, e intanto taglio i fondi agli enti locali, che quindi si ritrovano senza personale,

Stesso discorso per le Vepa e per le pergole bioclimatiche, che con questo nuovo testo saranno consentiti in edilizia libera. Lo sapete cosa vuol dire edilizia libera per queste tipologie di manufatti? Vuol dire volumi aggiuntivi senza alcun controllo. E ripeto: volumi aggiuntivi, perché le pergole bioclimatiche si chiudono completamente e fanno da tetto con i vetri; sono volumi aggiuntivi. Io lo dico, basta che si sappia. Introducete norme deregolatorie e non c'è un solo articolo, non c'è la minima traccia di risorse sul patrimonio edilizio pubblico. Lo voglio sottolineare, perché tutti abbiamo visto quanto è avvenuto tre giorni fa a Scampia: una tragedia che ci ha lasciati senza parole. La situazione in cui versano gli edifici residenziali pubblici in molte zone del Paese richiede attenzione e finanziamenti da parte dello Stato, per assicurare degne condizioni abitative. Portate in Aula un decreto casa che si occupa non del diritto all'abitare, ma solo di cancellare gli abusi edilizi. Concludo, signor Presidente, tornando a ribadire un concetto. Non si comprende l'urgenza di questo provvedimento. Non si capisce il motivo per il quale avete voluto cancellare il confronto, se non per i conflitti interni alla maggioranza. È un disegno di legge che aggiunge problemi e non risolve quelli esistenti. Avevamo davanti la possibilità di rafforzare il percorso di rigenerazione urbana e di semplificazione burocratica, anche e soprattutto mettendo le risorse per far lavorare bene i Comuni. Invece, avete scelto la strada della deregolamentazione, non della semplificazione, che serviva per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Nel mondo oggi il dibattito è tutto incentrato sulla sostenibilità, sulla conversione ecologica ed energetica. Voi vi presentate in Aula con delle norme che sembrano fuori dal tempo e fuori dalla storia, come se non avessimo conosciuto gli effetti dei condoni nel nostro Paese. Avete mostrato il pugno duro quando non serviva: contro i giovani con il decreto Caivano, con il decreto rave, con il disegno In questo caso, con i numeri drammatici degli abusi edilizi e l'illegalità che aumenta, vi risvegliate con una carezza. È per questo motivo che, a nome del Gruppo Partito Democratico, ribadisco la nostra totale contrarietà al voto di fiducia posto dal Governo.

Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, siamo oggi chiamati alla conversione del decreto che contiene misure urgenti per la semplificazione edilizia e l'urbanistica, che è stato enfaticamente chiamato dalla maggioranza di Governo decreto salva casa. Prima di entrare nel merito del provvedimento, io non mi rassegnerò mai a rivendicare la lesione delle prerogative del Parlamento. Visto che stiamo in un clima olimpico, direi che il Governo Meloni rischia di vincere la medaglia d'oro per il ricorso alla questione di fiducia con la decretazione d'urgenza: un primato di cui non c'è da essere orgogliosi. L'abuso della decretazione d'urgenza è ancora più problematico su questo provvedimento, perché comprimere il dibattito parlamentare su un tema così importante per tutti gli italiani come la casa penso sia irresponsabile. Il 70 per cento degli italiani è proprietario di casa. Modificare per l'ennesima volta la legislazione che riguarda la proprietà immobiliare significa dunque toccare la più grande voce del risparmio privato del nostro Paese: la casa. Ciò premesso nel metodo, nel merito il compito di chi, come Azione, svolge un'opposizione non ideologica è raccogliere la sfida di leggere e analizzare il provvedimento e dire ciò che di positivo e e ciò che di negativo c'è, cercando, attraverso la presentazione di emendamenti, di correggere gli errori nella prospettiva della riduzione del danno. Cosa c'è di buono in questo provvedimento? L'idea di semplificare la legislazione urbanistica per liberare gli italiani dal peso della burocrazia è giusta. Dirò di più: io trovo assolutamente giusto superare il principio della doppia conformità, ma vi pongo la seguente domanda. Se un proprietario di casa acquista una casa con un titolo legittimo e non fa alcun intervento di abuso edilizio, vi pare normale che poi non possa rivendere la sua casa perché, al momento del rogito, scopre di non riuscire a ottenere la relazione tecnica integrata perché manca la conformità rispetto al titolo vigente nel momento in cui è avvenuto l'abuso edilizio? È giusto superare il principio della doppia conformità per sbloccare il mercato immobiliare. Altro elemento positivo: bene il tema delle tolleranze costruttive, cioè la differenza tra quanto autorizzato e quanto effettivamente realizzato, in una soglia di tolleranza che arriva al 6 per cento per appartamenti non superiori ai 60 metri quadrati. Non è un condono: è una sanatoria edilizia che può sbloccare il mercato immobiliare, bloccato dalle piccole irregolarità con tramezzi e spostamenti di porte e verande. Ancora, noi giudichiamo positivamente la norma sul cambio di destinazione d'uso con una disciplina uniforme, senza distinzione, se con opera o senza. E allora cosa manca? non c'è in questo provvedimento che invece avrebbe dovuto esserci? Voi avete voluto chiamare questo provvedimento decreto salva casa. Ma se davvero aveste voluto salvare la casa agli italiani, avreste dovuto avere il coraggio di affrontare una tensione che cova nel nostro Paese e che si chiama emergenza abitativa. Ma qualcuno in quest'Aula pensa davvero che basti eliminare qualche laccio e lacciuolo del mercato immobiliare per risolvere il drammatico problema di chi una casa non ce l'ha o di chi una casa ce l'ha, ma non riesce più a mantenerla? Pensate che ai giovani e alle giovani coppie che cercano di acquistare una casa perché pagano un affitto che si mangia il 50 per cento del loro stipendio, noi possiamo rispondere con una norma sulle tende o sulle pergole bioclimatiche?

che non riescono più a mantenere la casa di proprietà e sono costrette a vendere tutto ciò che hanno per mantenere l'usufrutto dell'abitazione. E allora, se il problema drammatico è quello dell'emergenza abitativa, qual è la risposta? Non è questa che - come dicevo - al massimo è è una sanatoria edilizia. Voglio dire con chiarezza che per me la risposta non può essere neanche l'occupazione illegale. Non può essere questa la via per risolvere l'emergenza abitativa, né quando lo fa l'estrema sinistra, né quando lo fa a CasaPound. Quale sarebbe la via maestra? Sarebbe quella di un piano di investimento sulle case popolari, sull'edilizia residenziale, pubblica e privata. Non pensate che sia un problema solo italiano. La presidente von der Leyen, appena rieletta, ha detto chiaramente che una delle deleghe la prossima Commissione europea l'avrà sulla casa. La strada maestra che noi dobbiamo percorrere è il dovere di riqualificare il nostro patrimonio residenziale, pubblico e privato, sul tema dell'efficienza energetica, sul tema della sicurezza antisismica, sul tema della rimozione delle barriere architettoniche, fuori dalla logica dei *bonus*, ma con una politica industriale di lungo respiro. Dov'è tutto questo nel provvedimento? Non c'è. E allora chiamiamolo sanatoria edilizia, non chiamiamolo salva casa. Noi avevamo fatto proposte di emendamenti sul tema dei mutui per l'acquisto di prime case dei giovani, per gli studenti fuori sede, per gli alloggi popolari. Non li avete accolti e a proposito di ciò che manca e arrivo alla conclusione - non avete avuto il coraggio di accogliere una proposta su un tema, il salva Milano. Su questo il Parlamento ha perso una buona occasione di dimostrare coraggio e tempestività rispetto a un tema che sta bloccando le famiglie, gli investitori privati e i dipendenti del Comune di Milano, che si ritrovano con provvedimenti giudiziari emessi e pendenti sulle loro teste. Qui non si tratta di intervenire a gamba tesa in un conflitto tra la procura e il Comune di Milano. Si tratta di esercitare il nostro dovere costituzionale di fare chiarezza su un provvedimento legislativo ambiguo che crea incertezza per famiglie, investitori e amministratori pubblici. Avere rimandato a un prossimo decreto, probabilmente quello sulle infrastrutture, non fa l'altro che aggiungere ritardi e confusioni. Quello che manca, ed è il motivo per cui Azione voterà no alla fiducia a questo provvedimento, è una risposta strategica a un problema drammatico qual è l'emergenza abitativa. Difendere la rendita delle case dei piccoli proprietari, senza dare una risposta a chi non riesce più a mantenere la proprietà immobiliare e a chi non riesce a comprare una casa, è una scelta politica di corto respiro. Per questo Azione voterà contro la fiducia. *(Applausi)*.

pur sapendo che abbiamo probabilmente stessi obiettivi, ma strade diverse per poterli raggiungere. Mi sarei aspettato più facilmente magari una differenziazione tra chi ha avuto la fortuna di amministrare nei propri Comuni e chi non ha avuto una tale fortuna,

porre le basi di una piattaforma comune sulla quale poi intervenire per poter creare quello di cui effettivamente si avverte la necessità, ossia poter vivere

necessariamente intervenire per poter modificare e rendere agibili alcune situazioni che erano veramente drammatiche per alcune famiglie che si sono trovate nella disperazione più totale e più assoluta. però solamente agli utenti e ai proprietari degli immobili, ma anche ai tecnici comunali. I tecnici comunali si trovano nell'estrema e totale difficoltà di poter dare una risposta, perché non possono farlo secondo logica, non avendo un supporto normativo, quindi si trovano nella difficoltà di poter rilasciare un qualcosa che sembra evidente a tutti che possa essere rilasciato. Senza però un appoggio normativo non possono farlo. C'è il timore di andare

dando un termine al processo legato al superbonus al 110 per cento, ma non necessariamente chiudendo quello che è un adeguamento del dell'intero complesso edilizio nazionale, per poter raggiungere quell'efficientamento necessario e andare incontro all'evoluzione del sistema edilizio a livello generale. Questo provvedimento ha delle caratteristiche principali. Una è il superamento della doppia conformità, che veramente era diventata

in difformità a quello che era il progetto iniziale. Parliamo sempre del non uso di nuovo suolo quindi nuovo territorio, di mantenere l'edificato e poterlo sfruttare il più possibile: penso che questo consenta quantomeno di chiudere

per due mandati come assessore all'urbanistica. C'è tantissimo da lavorare, c'è tantissimo da fare, c'è eventualmente anche da togliere quel perimetro della città rispetto ai piani urbanistici, realizzando dei piani urbanistici con maggior respiro, lavorando su aree territoriali più vaste, in modo da creare effettivamente dei luoghi da poter vivere in maniera piena da parte dei cittadini, innalzando e qualificando le vocazioni di qualsiasi territorio. Quindi io penso che questa sia una base importante dalla quale ripartire per poter creare le condizioni per far sì che si possa lavorare per un miglioramento da un punto di vista edilizio e - questa volta sì - urbanistico del nostro Paese.

ma per noi rappresenta un punto di partenza che deve vedere il suo traguardo nelle nuove norme sulla rigenerazione urbana. infatti, lavorando su un ulteriore complesso di disposizioni che vedranno la rigenerazione al centro dello sviluppo delle città quale motore dell'edilizia e quindi dell'economia, di cui sono onorato di essere relatore in 8a Commissione. depositerò il testo unificato degli otto disegni di legge sulla rigenerazione urbana, quindi a breve in 8a Commissione potremo iniziare l'esame del provvedimento. Il decreto-legge al nostro esame ha il merito di avere nuovamente posto al centro dell'attenzione della politica il tema della casa e della necessità di mettere mano a norme vetuste che ne impediscono il pieno utilizzo e ne deprimono il valore. La casa è l'*asset* più importante degli italiani, posto che più di sette famiglie su dieci sono proprietarie dell'immobile in cui abitano. Per gli italiani la casa rappresenta il risparmio attraverso il quale si acquista un immobile per vivere, per i propri figli o per avere una fonte di reddito che vada a integrare la propria pensione; per gli italiani la casa rappresenta la storia della famiglia, le radici e lo stesso futuro della famiglia. Per gli italiani la casa rappresenta un sistema straordinario di *welfare*, costruito attraverso i sacrifici delle famiglie, che deve trovare una fonte di sicurezza nella normativa di riferimento. Si affianca a questi temi anche quello dell'emergenza abitativa, per chi ha difficoltà affrontare un mutuo, a trovare un alloggio compatibile con il proprio reddito. Il provvedimento in esame affronta queste tematiche mettendo al centro la necessità di soddisfare il crescente fabbisogno abitativo. La possibilità di sanare le irregolarità formali tutela la proprietà e amplia il numero di immobili disponibili sul mercato; allo stesso tempo, è l'occasione per recuperare una buona parte del nostro patrimonio edilizio, evitando un ulteriore consumo di suolo. inutile sottolineare che azioni di questo tipo, oltre a sostenere l'economia attivando il settore delle costruzioni e tutti gli altri settori economici collegati, muove il mercato immobiliare, lo sostiene e rappresenta una fonte di entrata ulteriore per lo Stato. Anche le amministrazioni pubbliche hanno chiesto di mettere in campo una grande opera di semplificazione, che inizia ora e che - ci tengo a ribadirlo - proseguirà nella legge sulla rigenerazione urbana. Gli uffici dei Comuni sanno quanto la complessità normativa rallenti l'azione amministrativa a fronte di strutture che, oltretutto, pagano spesso evidenti carenze di personale. il criterio seguito è stato quello di semplificare per recuperare immobili che oggi non potrebbero essere posti sul mercato. Gli interventi normativi riguardano il testo unico dell'edilizia, cui sono seguite le diverse disposizioni regionali in materia, che necessitava di essere integrato e modificato. Anche per queste ragioni il testo in esame deve quindi essere il punto di partenza anche di una nuova legge urbanistica, che dovrà avere un carattere organico, che valga sul territorio nazionale, che consenta le valorizzazioni e non le penalizzazioni attraverso la normativa regionale e locale. Si tratta di temi che coinvolgono anche la gestione del territorio e la prevenzione dei dissesti idrogeologici, che vanno coniugati con il bisogno di adottare necessarie trasformazioni urbanistiche. Si tratta di interventi non più differibili, posta anche la fragilità dell'intero territorio nazionale, già piegato dagli eventi naturali (ma che sono straordinari) degli ultimi anni. L'occasione è quindi propizia per dare il via a questa auspicata opera di razionalizzazione e semplificazione di tutta la normativa in materia. Allo stesso tempo, vanno introdotti strumenti di pianificazione più razionali, che partono dal recupero del patrimonio edilizio esistente, dalla messa in sicurezza del territorio e degli edifici, dalla sostenibilità energetica e ambientale, coniugando le esigenze dell'edilizia privata e residenziale con le necessità pubbliche. L'economia legata alla filiera delle costruzioni deve essere messa in grado di operare con tempi ragionevolmente veloci, con norme certe, di facile attuazione e che non inneschino inutili contenziosi tra il privato e il pubblico. Ecco quindi che proprio il completamento della normativa in esame, con il complesso di disposizioni previste dalla legge sulla rigenerazione urbana, potrà integrare quanto previsto da questo che già contiene molte disposizioni che intanto fanno fare un passo avanti al quadro normativo esistente. Ne elenco alcune. dal superamento della doppia conformità, anche per difformità sostanziali, posto che le leggi regionali trattano in modo diverso le parziali difformità edilizie, l'obiettivo è rendere più semplice e uniforme la sanatoria degli interventi edilizi. una norma per regolarizzare gli interventi edilizi eseguiti in parziale difformità rispetto al titolo, prima dell'introduzione del permesso di costruire, con una procedura semplificata per i titoli rilasciati prima del 1977. rende più facile e veloce il cambio di destinazione d'uso, rendendo uniforme la disciplina, con la possibilità di eseguire le opere previste in edilizia libera. Per determinare lo stato legittimo si farà riferimento all'ultimo titolo abilitativo rilasciato, fermo restando che spetta alle amministrazioni competenti verificare la legittimità dei titoli pregressi. Si introducono novità per le tolleranze degli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, per esempio per le unità immobiliari sotto i 60 metri quadrati sono tollerati scostamenti fino al 6 per cento e di questo vorrei ringraziare la Federazione degli agenti immobiliari per il vasto contributo di idee che ha dato al lavoro dei colleghi deputati, tra cui questa disposizione. la disposizione sui microappartamenti, per cui sarà possibile rilasciare il certificato di agibilità per abitazioni con superficie minima per una persona a 20 metri quadrati e per due persone a 28; c'è anche la possibilità di ridurre le Ovviamente tutto questo deve avvenire solo ed esclusivamente in edifici migliorati o ristrutturati per garantirne le idonee condizioni igienico-sanitarie. La norma agevolerà soprattutto studenti e lavoratori nelle grandi metropoli. Sarà più semplice il recupero dei sottotetti. Sono previste nuove categorie di interventi in edilizia libera, come la possibilità di realizzare vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti in tutti i porticati e l'installazione di strutture di protezione dal sole e dalle intemperie. Grazie all'approvazione di modifiche proposte da Forza Italia, i Comuni potranno utilizzare le somme derivanti dalla regolarizzazione delle difformità urbanistiche e dall'alienazione di immobili interessati da abusi anche per completare o demolire opere pubbliche incompiute oppure per aumentare l'offerta abitativa. Forza Italia da sempre ha posto la casa, il bene più prezioso degli italiani, al centro delle proprie politiche, lo hanno sempre dimostrato le politiche dei Governi Berlusconi. Ecco perché voteremo convintamente questo provvedimento, che risolve alcuni problemi urgenti in attesa di provvedimenti più corposi, come la rigenerazione urbana, che porterà a un nuovo modo di concepire le nostre città, tutelerà il valore degli immobili, rilancerà l'economia del settore dell'edilizia e del settore immobiliare, trasformerà le città in modo che siano più a misura d'uomo sotto il profilo sociale, culturale, del lavoro, della sicurezza, dei servizi e dell'ambiente. In sostanza, la rigenerazione urbana sarà una norma che disegnerà le città del futuro del nostro Paese.

come è emerso da questo dibattito (è la terza volta che intervengo sullo stesso tema), la nostra contrarietà a questo provvedimento è abbastanza chiara. E vorrei sottolineare che non è per niente pregiudiziale, anzi,

tecnici. C'è carenza di organico, tanto che c'è personale che lavora su più Comuni.

ma la casa in modo diffuso l'hanno costruita quelli che avevano un reddito fisso, perché su questo costruivano la casa. Io andavo in banca e questa mi concedeva il mutuo del fatto che sostanzialmente il mio reddito e quello della mia compagna garantivano questo prestito. Mia figlia, quando ha preso la casa, l'ha garantita suo padre, non lei, perché a un lavoratore precario non glielo danno il mutuo. Questo è quello che succede. Tante famiglie (cioè persone singole e persone coniugate o che abitano insieme) non hanno questa possibilità.

…non ne parla ed è per questa ragione che votiamo convintamente contro. Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, ormai la lettura in una delle due Camere è una formalità. E al Senato è talmente una formalità che, nel momento in cui almeno formalmente in quest'Aula

che vi sia un formale interessamento agli emendamenti presentati dalle opposizioni o agli ordini del giorno, anche perché, non essendoci il relatore, di fatto formalmente dovrebbe essere presente Presidente, per essere quello che ha depositato il verbo della maggioranza. Ormai anche la forma viene messa Sarà il caldo, sarà che siamo stanchi, saranno tante cose, ma ormai è proprio evidente che il bicameralismo è finito. E, visto che si mette mano alla Costituzione con il premierato, forse una riflessione in merito a un maggior funzionamento delle Camere sarebbe d'uopo. Fatta questa premessa sulla forma, che però è anche sostanza, veniamo a questo provvedimento, che - devo dire la verità - siete stati molto bravi a presentare come il piano casa. casa, infatti, riporta alla memoria il piano casa Fanfani, la Prima Repubblica, la ricostruzione dopo la guerra, l'avvio di un nuovo miracolo economico che vide protagonista il nostro Paese. Quindi, chiamarlo piano casa dava il segnale di qualcosa di estremamente positivo, rivoluzionario, che avrebbe fatto accelerare la produzione di nuova edilizia,

edifici e urbanistica. Anche lì, la parola urbanistica mi sembra eccessiva per quello che c'è all'interno del provvedimento, però poi, di fatto, si tratta di questo: di semplificazioni. Alcuni li hanno chiamati condoni: effettivamente, sono dei piccoli condoni a piccoli intoppi per quanto riguarda le costruzioni dei cittadini italiani. Intoppi che, in alcuni casi, non permettono la vendita

forse bisogna arrivare a una ridefinizione dei parametri edilizi piuttosto che prevedere ogni volta dei micro condoni. Quello che però è intollerabile è che questo Paese, in realtà, non ha bisogno di un provvedimento d'urgenza per piccoli intoppi degli appartamenti, perché non credo che tutti gli italiani vogliano vendere, in questo momento, case che abbiano delle manchevolezze. Quello di cui c'è bisogno, invece, è veramente di un piano casa: non dico come quello che fu di fanfaniana memoria, perché nel frattempo di case nel nostro Paese se ne sono costruite parecchie, ma perché ci sono sfide

A parte che, se non si è d'accordo, forse è meglio stare nelle stanze del potere e avere un commissario all'interno della nuova Commissione europea piuttosto che starne fuori; ma queste sono valutazioni politiche di questa maggioranza, che ha preferito starne fuori. Uno può essere anche non favorevole a quel provvedimento, ma quel provvedimento arriverà e forse bisogna costruire una modalità con la quale, ad esempio, sul nuovo verranno verranno individuati dei nuovi parametri di costruzione per prevedere come ristrutturare il vecchio: con che tempistiche, con che modalità, con che accesso al credito. Invece questo non viene fatto. Poi ci sono i vecchi problemi. L'edilizia pubblica è assente, con 600.000 famiglie che l'attendono, e non c'è abbastanza risorsa. C'è tutto il tema del mancato rifinanziamento del fondo sugli affitti di morosi non colpevoli. questo fondo manca dalla legge di bilancio e non è stato rimpinguato. Voi mi direte: ma noi governiamo da un anno e mezzo, chi veniva prima di noi doveva intervenire. Certo, ma c'è un piccolo dettaglio: soprattutto per quanto riguarda l'edilizia pubblica e l'edilizia che riguarda, per esempio, gli studenti universitari, voi avete i fondi del PNRR, cosa che i precedenti Governi non avevano. Quindi, avete un programma che dovrebbe sbloccare quei fondi, per arrivare ad una soluzione abitativa che interessi parecchie famiglie. Invece, voi decidete di fare in estrema urgenza,

C'è un tema che mi ha abbastanza colpito. Sulla parte urbanistica, in realtà, si prevede il silenzio assenso anche nelle zone di interesse paesaggistico. Mi è venuto un po' da sorridere. Infatti non più tardi della scorsa settimana noi abbiamo emanato il decreto agricoltura con il quale abbiamo bloccato il solare a terra, al grido di «salviamo i campi, salviamo l'agricoltura, prima il cibo e poi l'energia».

l'energia - il solare, l'eolico, tutto ciò che è rinnovabile - produce un depauperamento e deturpamento dell'ambiente e del paesaggio italiano, che è famoso in tutto il mondo e attrae turisti da tutto il mondo, che deve essere tutelato, e quindi le aree idonee sono molto stringenti. Infatti tra l'energia, le bollette degli italiani, la possibilità di dare un aiuto agli imprenditori che producono, eccetera eccetera, noi preferiamo il bello. Poi però arriva l'abuso edilizio e allora il paesaggio italiano diventa una delle tante cose che bisogna tutelare. Prima la casa, che è un diritto degli italiani, e quindi se c'è un bell'abuso edilizio del paesaggio, del turismo, delle colline, dei fiori e degli alberi non ce ne frega più niente. A quel punto facciamo non uno ma dieci passi indietro: silenzio assenso anche nelle zone vincolate. Mi sembra Mi sembra una tale ipocrisia che, diciamolo, questo Governo non vuole sbloccare il problema sull'energia, non gliene frega niente delle energie rinnovabili, spera di fare accordi in tutto il mondo per avere il gas di tutto il mondo, perché non vuole l'autosufficienza energetica

Questo non è un decreto casa, questo è un decreto che salva le irregolarità di alcuni italiani, con buona pace di chi ha rispettato le leggi che ancora una volta si vede assolutamente sbeffeggiato da chi invece dovrebbe tutelarlo, cioè lo Stato.

una delegazione degli amministratori della città di Cherasco, in provincia di Cuneo, rappresentati dal vice sindaco e dagli assessori

del ministro Salvini, che non ha ritenuto importante presenziare a questa discussione, come altri colleghi hanno sottolineato, siamo di fronte all'ennesima fiducia. In quest'Aula la discussione non è prevista. Il Parlamento viene relegato a un ruolo che definire marginale è sin troppo generoso e in linea con il futuro premierato che intende istituzionalizzare l'irrilevanza del Parlamento. Commissione, di cui sono membro, il tempo di discussione è stato praticamente inesistente: incardinato la mattina alle 11, durante la discussione in Commissione, alle ore 12,30, si fissava il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno alle ore 14,30 - considerate che la Commissione sarebbe proseguita per oltre un'ora - poi generosamente posticipato alle ore 15. Nessuna discussione degli emendamenti, perché non c'era tempo e quindi alle ore 19 il termine per il deposito degli emendamenti in Aula. Praticamente ci hanno detto: state zitti, perché quel che pensate non è di nostro interesse. Quindi riceviamo il provvedimento, come è arrivato dalla Camera. In realtà, quando è nato, questo provvedimento aveva anche qualche aspetto interessante, nel senso che una semplificazione era sicuramente dovuta, ma poi è stato trasformato dagli oltre 300 emendamenti di maggioranza presentati alla Camera ed ha assunto un connotato assolutamente diverso e non condivisibile. Dunque, fondamentalmente, si va ad incidere su normative esistenti a *spot*, anziché pensare di creare un approccio organico. Quindi, invece di agire in modo da creare un riferimento normativo omogeneo e sicuro, si interviene a *spot*, creando davvero un'estrema confusione - a questo punto, sì nell'interpretazione delle norme. Gli uffici tecnici comunali avranno seri problemi quando caleranno sui loro tavoli tutte queste pratiche. pratiche. Cosa accadrà, visto che è stato inserito anche il silenzio assenso? Non faranno in tempo a fare nulla, per cui qualsiasi domanda verrà automaticamente accolta. Come vogliamo definire una situazione di questo genere? È un condono! È un condono, licenziato sotto forma di semplificazione.

sono stati presentati dalle forze di maggioranza, ma non solo, e sicuramente non dal MoVimento 5 Stelle. Tali emendamenti sono stati ritirati in *corner*, perché evidentemente è subentrata la salvifica intercessione di qualche personaggio competente,

Viceversa, sarebbe stata dovuta la presentazione di un permesso per costruire. La differenza fondamentale è che, con il permesso di costruire è obbligatoria la creazione di un piano attuativo, che consideri

Milano è una città estremamente cementificata e con il caldo estivo si creano le isole di calore, che ne rendono la vivibilità insopportabile, paradossalmente soprattutto nelle ore notturne, quando l'asfalto e il cemento buttano fuori tutto il calore assorbito durante la giornata. Quindi, prevedere questi servizi a favore dei cittadini è fondamentale. Immaginiamo dove possono rifugiarsi un anziano o un'anziana a Milano, in piena estate, con un caldo incredibile: forse in un centro commerciale, passeggiando tra gli scaffali dei detersivi, alimentandosi di *hot dog* a basso costo? Non sarebbe forse preferibile avere

delle aree fosse stata fatta sulla base di tabelle, piuttosto che sul prezzo di mercato. Insomma, vi era tutta una serie di circostanze che andavano a ledere prima di tutto i diritti dei cittadini. Quindi sono ben lieta che questi emendamenti siano stati ritirati e confido che la maggioranza sia pervenuta a miglior ragione. Il ministro Salvini, che ha venduto sui *media* questo decreto-legge salva casa associato al decreto salva Milano, dice che li ripresenterà in altro decreto, forse quello infrastrutture. A mio A mio avviso, sarebbe bene che ci fossero un'attenta riflessione e una presa in considerazione degli aspetti che ho testé evidenziato. al merito di questo decreto-legge, manca totalmente quello che sarebbe servito, ossia una pianificazione strategica per l'offerta di alloggi

non viene assolutamente data una risposta. Circa l'emergenza del contrasto al dissesto idrogeologico e antisismico, si poteva pensare di prevedere qualcosa del genere. il recupero del patrimonio edilizio esistente. Il senatore Rosso, che è relatore nella mia Commissione degli otto disegni di legge sulla rigenerazione urbana - uno dei quali è mio - garantisce che prenderà in considerazione questi aspetti, considerando anche quello del consumo di suolo. Auspico che quantomeno in quella sede si riesca veramente a lavorare insieme, perché attualmente il consumo di suolo non è assolutamente arrestato: a Milano e soprattutto nel Nord Italia continua ad avanzare a un ritmo molto preoccupante, anche perché è una risorsa limitata e non rinnovabile, quindi andrebbe persa per sempre. Peraltro, in merito alla rigenerazione urbana, sono stati tagliati i fondi del PNRR e non si capisce bene

forse della campagna elettorale e, in secondo ordine, quella di cercare di salvare il famoso decreto Salvini salva Sala, cercando di portare a casa qualche risultato da quel punto di vista. Il MoVimento 5 Stelle è decisamente contrario a questo ennesimo pasticcio normativo che - ora sì - creerà grande confusione.

il Senato a esprimersi su una materia che siamo tutti d'accordo nel definire e considerare vitale. Parliamo della casa, quello che per gli italiani è il primo e più importante bene, infatti oltre il 70 per è possessore dell'abitazione in cui vive e continua comunque a ritenere che investire per avere un tetto sopra la testa sia la maggiore forma di sicurezza, anche personale. Ciononostante, in Italia esiste un'emergenza abitativa che riguarda le famiglie più povere, i più fragili e i giovani. Tra le motivazioni che ne stanno alla base non si può non citare la burocrazia e tutte le procedure di legge farraginose, lente e confusionarie che paralizzano oggi il settore. Regolamenti edilizi e piani regolatori dei Comuni spesso carenti oppure poco chiari o addirittura troppo rigidi hanno avuto nel tempo conseguenze deleterie proprio sull'aspetto abitativo

fastidi e pensieri ai proprietari, nonché danni economici perché, a causa di queste piccole difformità, tanti di loro non hanno potuto avere accesso agli incentivi o ai *bonus* messi in campo dallo Stato. Creano anche grossissimi problemi agli enti, che sono sovraccarichi di pratiche che non riescono a smaltire. Le difformità, infatti, incidono sulla commerciabilità degli immobili, quindi rappresentano un ostacolo, come già detto, alle compravendite e agli affitti, che vengono rallentati o del tutto bloccati, ingessando il mercato immobiliare e determinando, di conseguenza, anche una crescita dei prezzi sia delle case in vendita sia di quelle in locazione, a danno proprio delle famiglie meno abbienti o dei giovani che si affacciano al mondo del lavoro o degli studenti. Non dimentichiamo, in proposito, la recente protesta delle tende, ovviamente cavalcata strumentalmente in quell'occasione dall'opposizione. Certo, il testo unico per l'edilizia tuttora in vigore non aiuta, anzi forse è anch'esso parte del problema, a detta soprattutto degli addetti al settore: con i suoi ventuno anni di di operatività, è infatti una normativa ormai obsoleta e disallineata con le esigenze e le caratteristiche attuali del nostro patrimonio immobiliare, tanto che da più parti se ne invoca una riforma. Il ministro Salvini e questo Governo hanno dunque raccolto tutte queste istanze provenienti dai territori, dagli enti locali, dagli operatori del settore e dai cittadini stessi e sono intervenuti proprio per dare risposte e porre rimedio a questa situazione, semplificando la normativa e portando benefici su più fronti: per le famiglie, che saranno alleggerite dai fastidi burocratici, ma anche dai problemi economici; per la pubblica amministrazione, nella quale il funzionamento degli uffici sarà efficientato, alleggeriti dalla trattazione di migliaia di pratiche a questo punto diventate inutili. Avrà benefici anche il mercato immobiliare: infatti, velocizzando le pratiche e l'adeguamento delle piccole difformità, le compravendite e gli affitti saranno molto più facili, oltre che più numerosi, quindi ci sarà maggiore disponibilità di abitazioni da vendere e locare, con ripercussioni positive per chi cerca casa, ma anche sui prezzi, soprattutto delle locazioni che ovviamente, con più immobili offerti sul mercato,

l'abusivismo lo ha davvero praticato e lo sostiene evidentemente, come per esempio la parte più estrema della sinistra, che addirittura è arrivata a candidare e a far eleggere al Parlamento europeo una persona che si è macchiata del reato di occupazione abusiva della casa e che quindi ha pensato di usare questo reato come strumento per difendere difendere il diritto alla casa. *(Applausi)*. Noi, invece, per farlo abbiamo scelto, come sempre, la via della legalità, con norme che offrono una soluzione semplice e immediata alle piccole difformità, che riguardano piccole percentuali della superficie dell'immobile o la collocazione degli impianti o piccole aperture e così via, che oltretutto riguardano addirittura più della metà del patrimonio immobiliare italiano. Si tratta quindi di una soluzione che non intacca la sicurezza degli edifici, com'è stato sbandierato oggi in Aula, e che non disturba la quotidianità degli altri cittadini, ma evita ad esempio anche di consumare altro suolo, proteggendo quindi l'ambiente e la salute della collettività, determinando un grosso risultato anche sull'emergenza abitativa, come spiegavo prima. Per tutti questi aspetti, il provvedimento in esame avrebbe dovuto incontrare il favore assoluto di tutti i colleghi, innanzitutto della sinistra, che delle lotte per il diritto alla casa ha sempre fatto un suo baluardo. Citavo prima il movimento delle tende, rispetto al quale la sinistra si è schierata in prima linea per protestare contro il caro affitti per gli studenti; tuttavia, quando viene presentato un provvedimento che certamente non risolve il problema, ma può incidere in maniera determinante e positiva,

l'ipocrisia di chi si pone come paladino dei più deboli, ma solo a parole o, peggio ancora, perseguendo vie illecite o ancora suggerendo interventi contrari alla Costituzione che, ricordiamolo ancora una volta, tutela il diritto di proprietà come diritto fondamentale. Peraltro, voglio anche sottolineare come tutta una serie di interventi previsti dal decreto siano già operanti in altri Paesi europei, quelli governati dagli amici della sinistra e in quell'Europa che viene sempre portata ad esempio dai nostri detrattori magari proprio per criticare per criticare noi, la nostra azione e la nostra Italia. Mi riferisco ai microappartamenti, alla diminuzione delle altezze minime che altrove, come in Francia, sono addirittura inferiori a quella che ora noi prevediamo, o ancora al recupero dei sottotetti. Quello che evidentemente fa male all'opposizione è dover digerire che il ministro Salvini e il Governo di centrodestra stiano riuscendo a modernizzare finalmente l'Italia, a renderla efficiente e competitiva e a dare risposte ai cittadini che attendono da decenni nell'immobilismo e nell'incapacità proprio di chi ha governato finora fra continui no. *(Applausi)*. Noi invece, come diciamo, vogliamo essere l'Italia del sì, del vero progresso nell'interesse degli italiani, della sburocratizzazione e dell'innovazione che renda questo Paese competitivo, attraente e accogliente. Dunque anche oggi, a fronte di questo provvedimento, che riteniamo più che mai utile e benefico per tutti i nostri cittadini e che ha ricevuto, fra l'altro, il plauso delle Regioni, degli enti locali, di tutti gli operatori del settore e degli stessi cittadini, a nome del Gruppo Lega esprimo il convinto voto favorevole.

anche oggi ci troviamo a discutere di un provvedimento che solo per qualche ora questo ramo del Parlamento ha visto in Commissione, perché non ci è stata data la possibilità di discutere nessun emendamento. Anche oggi è arrivata una richiesta di fiducia

di fiducia è stata posta solo per questioni interne alla maggioranza, non certo per le opposizioni *(Applausi)*, che avevano anche offerto una disponibilità in Commissione a lavorare sugli emendamenti, in una discussione ampia. Non avete voluto, perché con la fiducia provate a risolvere le contraddizioni che iniziano a emergere all'interno della maggioranza. Avete battezzato questo decreto-legge salva casa. Noi pensiamo che potremmo ribattezzarlo salva abusi, perché sostanzialmente è nato male, nel Consiglio dei ministri, ed è finito peggio dopo il lavoro alla Camera dei deputati. Il Governo conferma un'enorme brama di potere: non riflette, non ascolta e si rifiuta di vedere. Si continua a mortificare il ruolo del Parlamento, a mostrare una grave intolleranza alla discussione e al confronto. Tra l'altro - ulteriore piccolo particolare - con un decreto di questo tipo, lanciato in pompa magna in campagna elettorale, che è stato approvato dalla Camera dei deputati, il ministro Salvini non si è degnato nemmeno di essere presente oggi né alla discussione generale, né alle dichiarazioni di voto, quando avrebbe avuto la possibilità di dire

sistema i problemi burocratici che da anni tengono in ostaggio milioni di famiglie italiane per qualche centimetro fuori posto, la finestra o la veranda, la mansarda o il sottotetto. Il Ministro, come al solito, minimizza, perché ha il vizio della semplificazione della realtà, se non dell'alterazione plateale. La verità è che questo decreto è un nuovo condono, è un provvedimento che non risolve l'emergenza abitativa e finisce per incentivare la speculazione edilizia a discapito dei più deboli, dei centri storici e dell'ambiente. Complimenti quindi al Governo, che rinuncia al popolamento dei centri storici, che, ad esempio, ignora le istanze degli studenti universitari e crea le condizioni per l'aumento degli affitti, altro che diminuzione dei prezzi, come veniva detto prima, peraltro in case di 20 metri quadri perfino senza aria. Tra l'altro, questo decreto va a modificare pesantemente il testo unico dell'edilizia, soprattutto rispetto alle norme relative alla legittimità degli immobili e alla loro regolamentazione. Anche Legambiente, in un rapporto di qualche mese fa, ci ha ricordato che l'annuncio di nuovi eventuali condoni alimenta l'illegalità. Anche i dati forniti dalle Forze dell'ordine ed elaborati nel rapporto ecomafia 2023 lasciano emergere che il ciclo del cemento illegale è stato nel 2022 il primo dei crimini ambientali accertati. Più volte abbiamo sottolineato che la casa è un'emergenza in Italia e le emergenze si affrontano con coscienza, preparazione, coraggio e ascolto. Vale per il tema della casa e, più in generale, per quello del governo del territorio. Invece il Governo crede che la soluzione individuata con questo decreto-legge sia rappresentata da alloggi di una sola stanza di 20 metri quadrati, ricavati in ambienti come cantine e sottotetti praticamente invivibili. Citiamo il dato dei 20 metri quadrati perché, consentendo alla svelta il cambio di destinazione d'uso di questi immobili, si favorirà la crescita di disuguaglianze e ingiustizie, perché darà spazio alla speculazione, agli affitti turistici e alla desertificazione delle aree urbane e storiche. Ne pagheranno le conseguenze i più poveri e gli studenti, che dovranno sopportare l'impennata dei canoni di locazione prodotta da speculazioni legittimate e incoraggiate da questo da questo L'emergenza e la precarietà abitativa rimangono un grande problema: finché esso resta senza una soluzione concreta, è inutile parlare di sviluppo economico, di politiche sociali e di misure per la famiglia. Per quanto riguarda l'agibilità, è stato modificato l'articolo 24 del testo unico dell'edilizia, autorizzando il progettista, in presenza di *standard* minimi, ad asseverare il progetto per i locali di altezza da 2,70 a

questa misura rimette sul mercato numerosi appartamenti, andando incontro a necessità di studenti e lavoratori, specialmente nelle grandi città, oltre a favorire la riduzione del consumo di suolo. Siamo al culmine della menzogna e dell'ipocrisia politica. Si permettono variazioni significative sugli immobili, anche di quelli sottoposti a vincolo o che ricadono all'interno di parchi e aree protetti sia nazionali sia regionali. Insomma, con un colpo di penna, si vanno a cancellare le norme più moderne di tutela del patrimonio storico e di salvaguardia ambientale. Tutto questo noi lo reputiamo scandaloso. Vengono inoltre sanate opere con significativi aumenti di cubatura, nonché difformi, realizzate in aree a rischio sismico. Stiamo discutendo in Commissione il decreto ricostruzione,

Eppure poi con norme urbanistiche di questo tipo creiamo un liberi tutti. Mettiamoci d'accordo: si può pensare di inseguire l'emergenza e poi dire invece di dove lavorare sulla prevenzione e, quando poi ci tocca lavorare sulla prevenzione, invece sull'altare della semplificazione si aggirano le norme, per esempio quelle antisismiche, in virtù di un decreto *spot* del ministro Salvini? Il provvedimento appare devastante e contiene ulteriori stravolgimenti delle norme di garanzia rispetto ai vincoli storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali e idrogeologici. In quanto al cambiamento della destinazione d'uso degli immobili, le modifiche che avete introdotto rischiano di limitare la possibilità dei Comuni di prevenire e arginare i fenomeni di degrado urbano. Bisognerebbe evitare la desertificazione dei centri storici, soprattutto a crescente pressione turistica, quindi la diffusione degli affitti brevi, spesso in residenze ricavate da fondi commerciali.

abbiamo provato a seguirne le indicazioni, inserendo correttivi in grado di salvaguardare gli strumenti urbanistici comunali. Purtroppo non c'è stato nulla da fare, a causa della miopia del Governo e della maggioranza e dell'impossibilità di discuterne anche in Commissione. Anzi, il centrodestra, di contro, ha dato il via libera a una *deregulation* assoluta. I Comuni sono scavalcati e messi in difficoltà. Se volevate semplificare, come avete provato a dire in tutti gli interventi della maggioranza, perché non aiutate i Comuni ad assumere personale qualificato per gli uffici tecnici comunali, che purtroppo ogni giorno vivono tra emergenze quotidiane, senza poter dare risposte ai cittadini? In sostanza, sono state cancellate tutte le regole sul cambio di destinazione d'uso; ne deriva che potrebbero essere stravolti interi quartieri delle città italiane. Altro che piccoli interventi di manutenzione. È un provvedimento assunto alla cieca, senza un confronto con le parti sociali, con la società civile e con le forze politiche, che alimenterà le disuguaglianze e colpirà gli inquilini, gli studenti fuori sede e le famiglie in difficoltà. Noi siamo fortemente contrari. Ma cosa sarebbe servito? Cosa serve al Paese? Cosa ci saremmo aspettati, dopo due anni di Governo? Probabilmente, la necessità di un salto di qualità, perché c'è il tema degli affitti, dell'acquisto, del recupero e della rigenerazione; c'è bisogno di un grande piano nazionale della casa, come ha proposto il Partito Democratico. Allora sarebbe stato corretto intervenire con uno specifico disegno di legge e discutere con le parti sociali attive nelle politiche della casa. Sarebbe servita una semplificazione normativa vera, preceduta da un'analisi dei fenomeni illegali che condizionano il mercato dell'edilizia. Questo si doveva fare, anche per non prestare il fianco ai furbetti dell'edilizia, in nome delle logiche e degli interessi di mercato. Bisognava semplificare il quadro normativo-legislativo riferito alle vecchie norme della pianificazione e dell'urbanistica, oltre a mettere mano, assieme alle Regioni, alla stratificata e contraddittoria legislazione regionale, che manda in tilt imprenditori, cittadini e professionisti.

una rigenerazione urbana non più rinviabile e dinamica, che riesca a interpretare i cambiamenti della società, delle città e dei cittadini, per un'urbanistica che riesca davvero a rispondere alle esigenze di un mondo e di una società che cambia. Lo dico sempre alla collega che sostiene che i corpi intermedi sono a favore di questo provvedimento. Qualche giorno fa ho partecipato a un'iniziativa dell'ANCE, in cui è stato presentato

ha fatto l'ANCE; lì c'è una grande voglia di discutere di rigenerazione urbana e non di un salva abusi. per due grandi cose che ha proposto: la prima è l'illusione di un ponte irrealizzabile (per il progetto che ha proposto); la seconda è questo condono di fatto, di cui il Paese non aveva bisogno e nemmeno i cittadini. Anche questa volta, il Governo si è girato dall'altra parte. Al salva abusi noi diciamo no. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo chiamati a votare in quest'Aula il decreto salva casa. Non il piano casa, ma il salva casa. Non il salva abusi, ma il salva casa. Il tema tocca da vicino la vita quotidiana di migliaia di concittadini. Il provvedimento origina dal decreto-legge n. 69, approvato dal Consiglio dei ministri il 24 maggio, su proposta del presidente Meloni e del ministro delle infrastrutture, il senatore Matteo Salvini. Ovviamente a loro va il ringraziamento corale, anche se, secondo una mia personale opinione, avremmo potuto e forse dovuto osare di più. Quando un territorio, nel caso nel caso specifico tutto il territorio nazionale, vive un disagio determinato da fattori vari, quali ad esempio il cosiddetto abuso di necessità, la politica ha il dovere di non girarsi dall'altra parte e di trovare soluzioni. Oggi sicuramente si compie un primo passo importante. Da ex sindaco di Bucciano, da uomo del territorio che mi vanto e onoro di essere tutt'oggi, ma anche quale segretario comunale, ho vissuto le difficoltà delle amministrazioni locali in questa delicata materia e mi sento in dovere di spiegare perché, per il centrodestra, questa non è solo una battaglia politica, ma una missione sociale. Voglio deludere subito chi dalla sinistra ci accusa di ogni male. Siamo qui oggi per difendere i diritti dei cittadini onesti, per offrire loro soluzioni concrete e per semplificare la loro vita, non certo per favorire gli speculatori edilizi. Il nostro impegno non è volto a promuovere sanatorie generalizzate, ma a risolvere piccole e complesse situazioni che affliggono i cittadini comuni, gli stessi che ogni giorno affrontano la burocrazia e purtroppo anche talune inefficienze dello Stato. È pleonastico, ma viste le posizioni di certa stampa e delle opposizioni, ritengo importante ribadire che questo provvedimento non è in alcuna maniera un condono edilizio che, come tutti sanno, è cosa diversa dalla sanatoria. uno strumento utile, essenziale, necessario ed urgente per risolvere in particolare le casistiche di minore gravità, snellendo le procedure e sburocratizzando il sistema, semplificando ad esempio la procedura della doppia conformità anche per le variazioni essenziali e introducendo il silenzio assenso in luogo del silenzio rigetto. È una misura a tutela della proprietà. Il cittadino, finalmente, potrà essere e sentirsi davvero proprietario, senza più vincoli e restrizioni burocratiche. A mio avviso, un punto fondamentale che consegue all'approvazione del provvedimento così come emendato alla Camera dei deputati è quello che tutela il legittimo affidamento dei proprietari che, avendo appunto legittimamente acquistato o realizzato immobili in assenza di irregolarità risultante da atti pubblici, si sono ritrovati nell'impossibilità di vendere i propri immobili, in forza di normativa sopravvenuta. Ancora, ai proprietari titolari di titoli edilizi non perfettamente validi per colpa dei Comuni, che, fino a una certa data, rilasciavano in zone vincolate concessioni edilizie senza aver acquisito preventivamente il parere obbligatorio delle competenti Sovrintendenze. Per dare una plastica rappresentazione dei miglioramenti conseguiti con il dibattito parlamentare, vi porto un esempio concreto, una testimonianza del nostro lavoro a favore della giustizia e della trasparenza. Alla Camera, come Fratelli d'Italia, grazie agli onorevoli Cangiano e Vietri e su mio impulso, abbiamo presentato un emendamento che è stato approvato e che, con poche righe, risolve, dopo decenni, una situazione catastrofica per molti cittadini, senza comportare oneri per lo Stato e che, anzi, garantirà solo introiti. Parliamo delle zone dove i cittadini hanno costruito, con regolare licenza edilizia e con regolare titolo edilizio, in aree vincolate, per le quali i Comuni, forse per un'errata interpretazione normativa, non avevano richiesto il necessario parere della locale Sovrintendenza. Questi cittadini si trovavano in un limbo burocratico da circa quarant'anni, bloccati da una mancanza amministrativa ad essi non imputabile. La soluzione di questo problema era stata sollecitata tantissime volte nel tempo. Da ultimo, a dicembre del 2023 tanti sindaci, della provincia di Benevento e Caserta, di ogni colore politico e di ogni parte d'Italia, i Presidenti di due Province e le Comunità montane, gli enti parco del Taburno e del Matese, gli ordini professionali, i corpi intermedi e le associazioni di categoria mi hanno sottoposto la questione ed hanno chiesto al Governo di dare una soluzione definitiva a questa problematica. Con il nostro emendamento, abbiamo posto fine a questa ingiustizia. Oggi questa proposta partorita nel Sannio è arrivata a Roma ed è stata inserita nel decreto-legge: una vittoria per chi ha duramente lavorato con determinazione e caparbietà, ma soprattutto per gli italiani e le loro abitazioni. Chi oggi, dalla sinistra dell'emiciclo, i dirimpettai, ci critica anche per questa soluzione, omette di dire oppure non sa cos'è successo in Emilia-Romagna. Con una legge regionale, la n. 24 del 2017, la Regione più rossa d'Italia da anni ha risolto la stessa problematica che oggi risolviamo noi con questo provvedimento a livello nazionale, eliminando un'inammissibile disparità di trattamento tra i cittadini italiani. Questo perché, evidentemente, quando si esce dal campo dell'ideologia e si vive il territorio, non si può negare che alcune battaglie siano giuste. quando la sinistra propone tali soluzioni, lo fa per nobili ragioni, per aiutare i cittadini in difficoltà. Se lo fa il centrodestra, siamo accusati di voler aiutare i furbi e gli speculatori. Questa ipocrisia è intollerabile e deve finire. È una narrazione distorta e pregiudizievole, che non tiene conto della realtà dei fatti. Noi siamo qui per aiutare i cittadini onesti, che rispettano le leggi e contribuiscono con il loro lavoro e i loro sacrifici. Non stiamo favorendo gli speculatori, stiamo cercando di offrire soluzioni reali a problemi reali per persone che si trovano in difficoltà, per colpa non loro ma di una burocrazia inefficiente e di normative confuse. Colleghi, dobbiamo combattere questa narrazione faziosa e agire con coraggio e determinazione, perché solo così potremo restituire fiducia e speranza a chi si sente abbandonato e inascoltato. Permettetemi allora di sottolineare un punto fondamentale: la destra deve avere il coraggio di fare la destra. *(Applausi)*. Una destra che piace alla sinistra non sarebbe tale e i cittadini ci hanno dato fiducia sapendo chi siamo e cosa rappresentiamo. Dobbiamo esserne orgogliosi: essere destra sociale significa anche credere in valori come la legalità, l'onestà e la responsabilità. Il diritto alla casa è sacrosanto, ma non si può tradurre nel diritto a occupare abusivamente una casa, così come piace a certa sinistra, quindi, al contrario di chi pensa che occupare le case di altri sia legittimo e si ispira al modello di chi oggi ci rappresenta in Europa, noi ci preoccupiamo di tutelare i cittadini che con sacrificio hanno acquistato una casa e vogliono finalmente sentirsi davvero proprietari. Si tratta di favorire il principio di legalità: se costruisci regolarmente una casa con il sudore della fronte e se, per sopravvenuta normativa, per la burocrazia non sei più in regola, lo Stato deve darti la possibilità di regolarizzare. Essere stato amministratore locale mi ha insegnato l'importanza di essere reali e concreti. Sappiamo che a Roma si deve discutere di grandi *dossier*, ma sappiamo anche che questi temi vanno affrontati con la consapevolezza che dietro ogni pratica ci sono persone, famiglie e storie di vita. Il nostro impegno è di risolvere e semplificare la vita di questi cittadini onesti e il decreto salva casa rappresenta un primo passo in questa direzione. Oggi abbiamo l'opportunità di dimostrare che siamo dalla parte dei cittadini. Votare a favore di questo decreto-legge significa dire sì a una politica che si preoccupa realmente delle persone, che agisce con responsabilità e guarda al futuro con fiducia. Continuiamo su questa strada insieme per un'Italia più giusta e solidale. Il centrodestra deve avere il coraggio di essere sé stesso. La casa per noi italiani è famiglia e convivialità, è serenità e stabilità. Per Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni la casa è sacra e con questo decreto la salvaguarda e la protegge. Dobbiamo agire con la forza delle nostre convinzioni, per il bene del nostro popolo e della nostra Nazione, consapevoli che finalmente stiamo cambiando l'Italia. Gli italiani possono stare tranquilli, difenderemo sempre le loro istanze e i loro diritti. Giorgia Meloni è al loro fianco e l'azione del nostro Governo punterà sempre più in alto, provando a risolvere le tante difficoltà ereditate e restituire stabilità e forza alla Nazione. Per questi motivi, annuncio il voto favorevole al provvedimento e quindi la fiducia al Governo Meloni del Gruppo Fratelli d'Italia.

nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione

senatrice Segretaria dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza. I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge

Signor Presidente, permettetemi di esprimere nuovamente il cordoglio ai familiari delle vittime del crollo di Scampia. L'intervento di oggi è volto ad affrontare una questione anch'essa di estrema urgenza e importanza per la nostra comunità: la violenza nel mio comune di Torre Annunziata. Venerdì scorso, in un ambiente che dovrebbe essere sicuro e gioioso, come una spiaggia, abbiamo assistito a un atto inaudito di violenza: due uomini a volto coperto hanno aperto il fuoco in un affollato lido, seminando il panico e il terrore tra i bagnanti. Questa aggressione non è un episodio isolato, ma rappresenta un'inquietante tendenza che colpisce la nostra realtà quotidiana. Io desidero esprimere il mio riconoscimento alle Forze dell'ordine perché si sono prontamente attivate e ringrazio anche il prefetto di Napoli, dottor Michele Di Bari, che ha risposto prontamente convocando il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. È fondamentale che tale attenzione venga mantenuta alta. Onorevoli colleghi, la presenza di quei criminali armati è inaccettabile, soprattutto in un luogo come una spiaggia. È nostro dovere garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire che simili episodi possano ripetersi. La situazione richiede un intervento coordinato, che preveda non solo un rafforzamento delle Forze dell'ordine, ma anche iniziative concrete di supporto per le istituzioni locali e per la comunità. In questo contesto sollecito un intervento robusto e deciso da parte del Governo. Non basta focalizzarsi su un caso - penso a Caivano - ma è necessario adottare strategie globali che affrontino la criminalità in tutte le sue forme, non solo nelle aree più visibili. Ho ripetutamente sollecitato, anche attraverso un'attività emendativa sempre respinta da questa maggioranza, l'aumento delle risorse destinate alla sicurezza e al potenziamento delle Forze di polizia, in particolare del Corpo di polizia municipale, che è sotto organico. Propongo anche di investire nella rinascita economica della nostra zona, integrando lavoratori in difficoltà nel nuovo *hub* turistico commerciale Maximall di Torre Annunziata. Questo approccio non solo favorirebbe l'occupazione, ma contribuirebbe anche a creare un clima di sicurezza necessario per attrarre investimenti. Auspico che le istanze che porto avanti non cadano nel vuoto. È urgente che l'Esecutivo attui una strategia di prevenzione efficace. La sicurezza non è solo un obbligo etico, ma è anche un elemento chiave per lo sviluppo economico. Concludendo, sottolineo l'importanza di un maggiore presidio delle Forze dell'ordine a Torre Annunziata. Dobbiamo garantire pattugliamenti costanti, in particolare nelle aree più a rischio. Ogni cittadino deve potersi sentire sicuro, libero dalla paura. La bellezza della libertà richiede un'azione collettiva. Onorevoli colleghi, signori del Governo, non lasciateci soli.